L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Il decreto-legge era composto inizialmente da 51 articoli e, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, risulta ora contenere 96 articoli suddivisi in quattro Titoli. Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 15, reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 e si compone di sei Capi. Il Capo I, dall'articolo 1 all'articolo 4, 4, detta disposizioni in materia di turismo. L'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo, fieristico e congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto. L'articolo 2, invece, utilizzando i fondi previsti dal PNRR, istituisce nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale turismo per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i turistici e i parchi tematici. L'articolo 3 prevede contributi alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, mentre l'articolo 3-*bis* Il Capo II, che va dall'articolo 5 all'articolo 6-*quater*, detta disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche. L'articolo 5 modifica le procedure di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI (Rete ferroviaria italiana). L'articolo 6 detta norme volte ad accelerare i tempi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e dispone misure in materia di edilizia giudiziaria. L'articolo 6-*bis* introduce alcune disposizioni volte a promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche. L'articolo 6-*ter* riscrive la disciplina sugli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. 6-*quater* riguarda i compensi dei collegi consultivi tecnici delle stazioni appaltanti. Il Capo III, composto dal solo articolo 7, detta disposizioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Il Capo IV, che va dagli articoli 8 al 10-*bis*, detta disposizioni relative alle procedure di spesa e controllo parlamentare. Si segnala l'articolo 9 che detta norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento - credo che sia importante sottolinearlo nel processo di attuazione e valutazione delle spese del PNRR. Il Capo V detta disposizioni in materia di zone economiche speciali (ZES), prevedendo all'articolo 11 lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle zone economiche speciali, nonché semplificazioni procedurali per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza dei servizi. Il Capo VI, che va dall'articolo 12 al 15, detta disposizioni in materia di università e ricerca. L'articolo 12, in particolare, semplifica i requisiti di eleggibilità per l'accesso da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre l'articolo 13 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. L'articolo 14 stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che una parte dei crediti formativi universitari può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, con l'obiettivo di semplificare le procedure e di favorire il rispetto di elevati *standard* ambientali. Il Titolo II, composto dagli articoli che vanno dal 16 al 40, reca ulteriori misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR e si compone di cinque Capi. Il Capo I, dagli articoli 16 al 19-*ter*, detta disposizioni in materia di ambiente. In particolare l'articolo 16 reca varie norme in materia di risorse idriche, mentre il 16-*bis* proroga di due anni l'affidamento del servizio idrico integrato alla Società acquedotto pugliese SpA. L'articolo 16-*ter* prevede una disciplina di accompagnamento all'apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica. L'articolo 17 prevede l'adozione da parte del Ministero della transizione ecologica di un piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinanti orfani, attuativo delle previsioni del PNRR. L'articolo 17-*bis* prevede l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e per la riperimetrazione dei siti contaminati e attualmente classificati di interesse nazionale (SIN). L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale (VAS). L'articolo 18-*bis* reca modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. L'articolo 19 reca disposizioni in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, mentre il 19-*bis* modifica la disciplina degli impianti a fonti rinnovabili, beneficiari di incentivi più risalenti (Certificati verdi, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio). L'articolo 19-*ter* disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo da parte di commercianti e professionisti di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto di pagamento di qualsiasi importo. concerne gli articoli dal 20 al 23, detta disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di coesione territoriale. l'articolo 20 introduce norme relative all'attribuzione di contributi statali ai Comuni in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, messa in sicurezza e valorizzazione del 20-*bis* detta norme volte alla semplificazione e all'accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 avvenuti in Abruzzo. L'articolo 21 dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane, mentre il 22 disciplina l'assegnazione delle risorse previste dal PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. L'articolo 23 consente l'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020. Il Capo III, del Titolo II, detta disposizioni in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari. L'articolo 24 demanda al Ministero dell'istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, mentre il 24-*bis* stabilisce che a partire dall'anno scolastico 2025-2026 nelle scuole di ogni ordine e grado si prosegua lo sviluppo delle competenze digitali. L'articolo 25 prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020. L'articolo 25-*bis* reca disposizioni relative alle attività della ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR.

la pandemia ha mietuto oltre 5,5 milioni di vittime nel mondo, provocando lutti, sofferenze e paure. La gravissima crisi che ha accompagnato l'incedere inarrestabile rapida diffusione del *virus* ha reso indispensabili scelte difficili, estreme e anche impopolari, ma che, nell'attesa che la campagna vaccinale decollasse e rappresentasse un argine alla diffusione del *virus* e un'ancora di salvezza cui affidare la nostra vita, ci hanno permesso di arrivare a questo punto. Le scelte fatte dal Governo Conte II, prima, e poi confermate dal Governo Draghi, che le ha ulteriormente potenziate e modulate in rapporto al variare delle condizioni epidemiologiche, hanno fatto dell'Italia uno dei punti - se non il punto - di riferimento per gli altri Paesi europei che, pur partendo da posizioni differenti, hanno adottato misure e provvedimenti simili a quelli presi dall'Italia. L'enorme sforzo economico dell'Europa, con la pioggia di miliardi di euro che ogni Stato membro ha ricevuto, ha presupposto l'elaborazione di piani strategici programmatici che consentissero, in un primo momento, di far fronte e resistere alla crisi globale provocata dalla pandemia e, successivamente, permettessero la ripresa e un vero e proprio scatto in avanti. Gli ingenti fondi ottenuti dall'Unione europea dal presidente Conte costituiscono la base finanziaria indispensabile che sostiene il Piano nazionale di ripresa i suoi progetti e missioni, che dovranno consentire al nostro Paese, dopo la fase emergenziale, di riprendere, come tutti noi ci auguriamo, una crescita globale non solo delle attività economiche e dell'occupazione, ma anche permettere un cambiamento radicale della nostra strutturazione e un ammodernamento tecnologico e delle infrastrutture. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, l'importanza della realizzazione, prevista dalle varie missioni del PNRR, di politiche attive, di coesione e inclusione: la rivoluzione verde e la transizione ecologica, la transizione digitale e la riorganizzazione del nostro servizio sanitario. È fondamentale e indispensabile che il cronoprogramma previsto dal PNRR sia rispettato nei tempi e nelle modalità. I vari progetti che si ricollegano alle sei missioni del Piano sono destinati - nelle intenzioni e, speriamo, nella loro realizzazione - a contribuire a quel cambiamento radicale e a quello scatto in avanti del nostro Paese che permettano all'Italia di allinearsi, non a parole, ma nei fatti, ai Paesi *leader* europei. È un momento importante, che coinvolge tutti gli aspetti, le attività e i delicati equilibri della nostra collettività, permettendo una sua graduale ma profonda modernizzazione. Signor Presidente, non dobbiamo dimenticare, tra le missioni previste, l'attenzione mostrata a investimenti programmati per il sostegno alle persone fragili

a rafforzare l'autonomia delle persone disabili e il loro inserimento sociale e lavorativo. La prevista riorganizzazione sanitaria comporterà, da un lato, il potenziamento della medicina territoriale (con integrazione tra i servizi sanitari e sociali e la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità) e, dall'altro, piani di riorganizzazione e ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

l'adozione delle modalità per l'istituzione del Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali e l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* di genomica estesa (Next Generation Entrambi avranno un ruolo fondamentale per le patologie oncologiche e il loro approccio terapeutico. Fondamentale per il rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR è la presenza della cabina di regia centrale, con compiti di supervisione, di indirizzo, di impulso e di coordinamento generale nell'attuazione degli interventi previsti, oltre che di ricognizioni periodiche e puntuali sullo stato di attuazione dei progetti, sulla loro efficacia e sul loro impatto rispetto agli obiettivi perseguiti. In parole povere, signor Presidente, essa deve poter svolgere un ruolo di controllo affinché i finanziamenti previsti siano spesi bene, nell'interesse dei cittadini e delle comunità, e vigilare affinché questo enorme flusso di denaro pubblico segua in maniera corretta i canali previsti e non possa richiamare gli appetiti mai sazi di organizzazioni malavitose, mafiose mafiose o camorristiche che siano. Qualora tali incresciosi episodi si dovessero verificare, occorre contrastarli, combatterli in maniera ferma e decisa e ribadire con forza la presenza dello Stato. Occorre correre, fare uno sforzo supplementare, ma fare le cose per bene, nell'interesse della collettività e non di singoli soggetti o *lobby*, recuperando i *target* e gli obiettivi previsti, anche quelli che attualmente sono in ritardo. il coinvolgimento del Parlamento è fondamentale in questo cammino di crescita e di programmazione, riconoscendo la sua centralità, d'altronde sancita dalla nostra Costituzione. Il MoVimento 5 Stelle c'è, sarà vigile, un controllore costruttivo, attivo, attento alla corretta attuazione del PNRR. Lo dobbiamo per rispetto a tutti i cittadini e, mi permetta, signor Presidente, come ricordo dovuto e sentito delle decine di migliaia di vittime della pandemia. *(Applausi)*.

rappresentanti del Governo, ci sarebbero molte cose da dire sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mi limiterò a fare qualche riflessione, cercando di contestualizzarla all'interno delle dinamiche politiche delle ultime ventiquattr'ore, provando poi a fare qualche altra considerazione di carattere tecnico-politico sul settore del turismo e sulla digitalizzazione. Il *premier* Draghi, quando presentò il Piano a quest'Assemblea, disse che l'Italia con esso avrebbe dovuto combinare l'immaginazione, la capacità progettuale e il pragmatismo. Questo per poter consegnare alle future generazioni, un Paese molto più moderno all'interno di un contesto europeo, che deve contare di più a livello mondiale e che deve essere molto più forte e solidale. La descrizione sintetica di questo Piano da parte del *premier* ci fa chiaramente capire che è l'occasione storica per il nostro Paese per superare una serie di indicatori che hanno caratterizzato i primi vent'anni del XXI secolo, che poi andrò a breve e che, secondo me, noi tutti dovremmo avere molto chiari nella nostra testa. Si tratta di indicatori che non possiamo assolutamente dimenticare in termini in termini economici e sociali e dai quali dobbiamo partire per determinare le condizioni di crescita e sviluppo di questo secolo. Ciò che il *Premier* ha riferito ieri,

tutto quello che ha fatto il Governo fino adesso è più che sufficiente per creare le condizioni per attuare questo Piano a nostro personale avviso - credo di poter parlare a nome dei colleghi di Forza Italia convincente. Certo, è stato fatto molto sul piano delle vaccinazioni, sono stati rispettati i termini per consegnare il Piano, l'Italia è cresciuta più delle previsioni (siamo al 6 per cento di crescita del PIL), però tutto questo non è assolutamente sufficiente. Peraltro, il *Premier* stesso ha detto che le persone sono importanti. Mi verrebbe da dire che le persone fanno la differenza, fanno il successo o l'insuccesso di un determinato progetto. Quindi, per ritornare a parlare del Piano, noi riteniamo che il *premier* Draghi debba effettivamente adoperarsi per calarlo a terra. È chiaro che lui da solo non basta, ci vuole una grande concertazione da parte di tutte le istituzioni: mi riferisco al Governo, al Parlamento, alle Regioni e a tutti gli enti locali. una concertazione sul piano istituzionale che sicuramente è molto complessa, ma che va assolutamente portata avanti per l'ambiziosità dei contenuti di questo Piano, per dargli dargli concreta attuazione e dunque consegnare - riprendo le parole che ho detto all'inizio - alle future generazioni un Paese completamente diverso. è sicuramente qualcosa di più complesso rispetto a qualsiasi evento internazionale, sia esso un'Olimpiade o un'Expo; lo dico perché recentemente ho sentito il sindaco Sala Sala dire che Milano deve dare un segnale a livello nazionale e deve fare qualcosa di estremamente importante, esattamente come ha fatto in occasione dell'Expo del 2015.

deve ritornare alla logica della programmazione (se non vogliamo utilizzare il termine "pianificazione" che forse è un po' forte e di natura bolscevica) e dobbiamo ritornare a programmare, esattamente come facevamo negli anni Sessanta, quando la programmazione costituì la novità nella gestione dello Stato. Oggi questa programmazione consentirebbe di andare oltre determinati numeri, che mi piacerebbe ricordare: tra il 1999 e il 2019, il PIL dell'Italia è cresciuto del 7,9 per cento e, nello stesso periodo, in Germania, in Francia e in Spagna l'aumento è stato rispettivamente del 30, del 32 e del 44

quelli che non studiano e non sono occupati, è significativamente più alto rispetto alla media europea; allo stesso modo, il numero di donne che partecipano attivamente al mondo del lavoro è significativamente inferiore rispetto alla media europea. la produttività, cioè il PIL per ora lavorata, tra il 1999 e il 2019 è cresciuto del 4,2 per cento in Italia, a fronte di un 21 per cento circa di Germania e Francia. Tra le cause di questi indicatori, che sono drammatici e che credo tutti noi dovremmo avere molto chiari nella nostra testa, per raccontarci che cosa è successo nei primi vent'anni di questo XXI secolo e per essere veramente convinti che ci vuole forte discontinuità da ora in avanti, dobbiamo ricordare sicuramente il fatto che la rivoluzione digitale non è stata compresa dalla politica industriale di questo Paese, così come la caratteristica del tessuto produttivo italiano, il cosiddetto nanismo, cioè le piccole-medie imprese e le micro-piccole e medie imprese, che sono anche la spina dorsale del nostro Paese e alle quali questa rivoluzione digitale deve prestare una grande attenzione. cosa dobbiamo fare con questo piano? Dobbiamo impostare una nuova politica industriale, dove la presenza dello Stato diventa centrale, non solo per rilanciare l'economia, ma anche per gestire i cosiddetti capitali pazienti, quelli di medio-lungo termine, quelli per i quali - si dice così - il *payback*, il ritorno non è assolutamente pensabile possa essere accettato dai capitalisti privati. Il PNRR deve sostanzialmente essere considerato - per riutilizzare delle parole del presidente Draghi - come una leva straordinaria una leva straordinaria che attira i capitali privati in una *partnership* virtuosa pubblico-privato che rilanci la nostra economia. Se così non fosse, l'Italia perderebbe l'occasione storica di questo secolo e la crescita di sviluppo del nostro Paese rispetto a quella degli altri Paesi europei diventerebbe così larga da portarci in una posizione di isolamento. Possiamo dire oggi che, dopo la pandemia, siamo tutti ai nastri di partenza e da qui inizia la gara, che non iniziamo con una penalizzazione perché sappiamo che la Commissione europea

la capacità di calare a terra questo Piano. Vado all'ultima considerazione, quella sul turismo. Spero che il ministro Garavaglia, che abbiamo peraltro convocato in 10a Commissione, venga a spiegarci, proprio perché sul turismo la digitalizzazione svolgerà un ruolo estremamente importante, che cosa è questo *hub* nazionale del turismo. Spero che sia un nodo dell'ecosistema digitale attorno

un contributo significativo in termini di crescita del PIL del comparto. Su quel comparto, che non è solo turismo ma è anche il meglio del *made in Italy*, penso che il nostro Paese possa fare dei punti di crescita di PIL significativamente importanti, quelli che non ci sono stati nei primi vent'anni, nonostante il settore non soffrisse, come molti possono constatare guardando i numeri. Vi è però un potenziale inespresso che deve assolutamente emergere e può essere valorizzato attraverso questo modo di fare politica industriale, che sia di riferimento per il comparto del turismo.

termali, i porti turistici, i parchi tematici, fieristici e congressuali. Su cosa in particolare si va a concentrare questo tipo di misura? Sull'efficienza energetica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi edilizi, interventi per la realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature funzionali alle piscine termali, gli interventi di digitalizzazione del comparto. In favore di questa misura sono stanziati ben 500 milioni Oltretutto, è stato inserito alla Camera durante la prima lettura - ormai di lettura se ne fa una sola quindi oggi prendiamo atto che alla Camera hanno fatto un buon lavoro - un fondo di 10 milioni di euro a fondo perduto per quelle imprese del settore della ristorazione che tanto si sono trovate in difficoltà in questo periodo pandemico. Ci sono poi garanzie sui finanziamenti del settore del turismo, un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

un incremento, anch'esso disposto alla Camera, di ulteriori 100 milioni per il fondo sul turismo. Esiste un credito d'imposta per un altro settore del comparto molto messo in difficoltà,

che non è più un di cui, di qualcos'altro o di qualcun altro, ma un Dicastero con una sua dignità: finalmente qualcuno può battere i pugni sul tavolo del Consiglio dei ministri per dire che esiste un comparto che fa 13 punti di PIL che si chiama turismo, all'interno del quale ci sono imprese

che riempie il cuore, dà fiducia e speranza - anzi, direi ottimismo - perché non so se parlare di speranza in questo momento porti così tanto bene, in realtà. In quest'ottica, le risorse del PNRR sono fondamentali.

in montagna o nelle nostre città d'arte o fare il percorso dei nostri piccoli borghi, quella miriade di posti fantastici pieni di cultura e di tradizione

Come si diceva, tutto il lavoro che è stato svolto fino ad oggi e probabilmente quello che si svolgerà successivamente è fondamentale per la sopravvivenza di questo comparto, che ha subito davvero un colpo quasi mortale. Chi, come me, viene da una famiglia di commercianti non può che provare a esortare questo Governo ad aumentare davvero gli sforzi per il commercio, specie per i piccoli negozi, la piccola ristorazione, trecentosessantacinque giorni all'anno, con ogni clima, con ogni avversità e - mi viene da dire - con ogni pandemia, tengono vivo un tessuto sociale fatto di servizi.

e città e l'abitudine di andare al ristorante o dal nostro commerciante di fiducia verrebbe meno. Non vorrei che tutto si tramutasse in un *click*, che mi sembra la cosa peggiore che ci possa capitare. Concludo con una riflessione che mi sta molto a cuore, su quello che sta accadendo alle 30.000 imprese italiane del settore balneare. Una sentenza del Consiglio di Stato

La politica, che è stata più volte richiamata ad assumersi le proprie responsabilità - voglio far presente che si sono succeduti tanti Governi, da quando si è posta la questione balneare - in realtà con la legge n. 145 del 2018, che disegnava un percorso, concordato con l'Europa, che avrebbe messo in sicurezza quelle 30.000 imprese e le loro famiglie.

rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è fondamentale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che non è solo il piano nazionale di questo Governo, ma è il piano di rilancio di tutto il nostro Paese spetta quindi a tutti noi - politici, funzionari, imprenditori e parti sociali - contribuire alla sua giusta realizzazione, in modo rapido ed efficiente. infatti che abbiamo solo cinque anni per investire in Italia 191,5 miliardi di euro e dobbiamo investirli nel modo giusto, con progetti che siano ecosostenibili. Tali fondi serviranno quindi a ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere e quindi ad accelerare la transizione, sia digitale sia ecologica, ma anche a migliorare la scuola, a rafforzare la sanità, a riformare in modo profondo l'economia e quel modello economico che probabilmente finora forse ha fallito, a rilanciare la produttività, a semplificare la burocrazia, a favorire l'innovazione e a diminuire la disoccupazione e dare lavoro ai nostri giovani, perché restino in Italia. Nel provvedimento in esame ci sono diverse norme che riguardano il Sud e anche il mio territorio, la Puglia, con tematiche di tipo ambientale. Ricordo ad esempio l'articolo 16-*bis*, che proroga di due anni l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese SpA. Tale proroga è stata introdotta «al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo

che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, Un altro importante passo avanti è stato fatto con l'articolo 17, che riguarda i siti orfani. A tale proposito, ricordo il lavoro costante che è stato fatto dal nostro ministro Costa su questo punto particolare.

e anche per i veicoli fuori uso e le pile. Nel 2019, la raccolta differenziata dei RAEE è stata del 39 per cento rispetto all'immesso e al consumo, percentuale ben lontana da quel del 65 per cento del *target* europeo. Stesso discorso vale per i veicoli fuori uso, la cui percentuale di impiego e riciclo, rimane lontana dal 95 previsto per i prossimi anni. La causa principale è la difficoltà di trattamento di alcuni componenti dei veicoli,

ultimi sono per noi importanti, perché dobbiamo migliorare l'efficientamento energetico, la rigenerazione urbana, la messa in sicurezza e la valorizzazione del territorio, la mobilità sostenibile e in particolare in particolare anche la messa in sicurezza delle nostre scuole, degli edifici comunali e del patrimonio comunale, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche. A tale riguardo, ricordo che già nel 2020 è stato assegnato un importo pari a 497,22 milioni di euro.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede di rivitalizzare e migliorare le grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi per la persona e la riqualificazione

I nostri nuclei urbani non devono essere più pensati come un conglomerato di individui, ma anche come laboratori di innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile. All'articolo All'articolo 50 si parla del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria. Sono quindi necessari investimenti per la riconversione delle imprese verso modelli di produzione sostenibili e la promozione della bioeconomia e dell'economia circolare.

Signor Presidente, colleghi, Governo, il decreto-legge che ci apprestiamo a votare oggi in Aula è essenziale e funzionale a imprimere un'ulteriore e decisiva spinta alle riforme e agli investimenti del PNRR. Siamo peraltro prossimi alla prima scadenza di verifica, che sarà il 31 dicembre,

Alla ripresa, a gennaio, proprio qui in Senato si aprirà la fase della verifica, per capire come si è arrivati a raggiungere questi obiettivi e come l'impegno straordinario di questi mesi abbia consentito all'Italia di essere tra i primi Paesi europei in fatto di crescita

si interviene sull'attuazione del PNRR, dal momento che contiene diverse e importanti misure, che toccano svariati temi e settori. Qualche collega prima di me ha citato opportunamente il turismo, che è un architrave del modello di sviluppo di questo Paese. Ci sono misure importanti, che toccano anche l'accelerazione delle iniziative in materia di ambiente, efficientamento energetico e rigenerazione.

ragionarci un po' di più anche qui in Senato. Il tempo è - ahimè - stringente e abbiamo dimostrato che il legislatore italiano è tutt'altro che inerte. Nelle prossime settimane, il nostro contributo sarà quello di verificare in concreto l'attuazione del PNRR, per misurare il tasso di raggiungimento degli obiettivi,

è qualcosa di diverso rispetto agli strumenti con i quali ci siamo confrontati in quest'ultimo ventennio. È il primo strumento di politiche fiscali comuni attraverso il quale si raggiungono - o si devono raggiungere - specifici risultati quantificabili, che saranno misurati dalla Commissione europea, e solo al positivo raggiungimento dei *target* progressivi saranno erogate le rate successive. È un cambio di mentalità importante, perché non solo l'Europa raccoglie le risorse e le redistribuisce, ma ci indica gli obiettivi da raggiungere e ci impegna a traguardarli. Voglio dire

forse mi tiene in una posizione diversa rispetto ad alcune rivendicazioni, perché credo che in questo strumento la regia nazionale sia un fatto importante. Dico questo Dico questo per provare a controbattere garbatamente all'intervento di qualche collega che ho sentito ieri in Aula. Si parlava di bilancio, ma siamo andati a riflettere anche sul PNRR. La regia nazionale ci serve per provare a risolvere finalmente una serie di divari territoriali che condannano questo Paese a una velocità inferiore alle sue potenzialità.

sanità diverse da altri territori di questo stesso Paese. Credo che la regia nazionale debba aiutarci a conseguire il traguardo di assicurare diritti universali al Sud come al Nord, con gli stessi *standard* e con le stesse possibilità di usufruirne. Vi dico che su questo continuerò a dare battaglia con ogni energia, perché è finito il tempo di immaginare che, se al Sud non si può contare su un sistema sanitario all'altezza delle necessità, è colpa del presidente di Regione di turno. Penso che lo Stato debba tornare a fare lo Stato e uno Stato

prodotto sin qui risultati molto al di sotto delle attese e abbiamo tutta una serie di misure attraverso le quali dobbiamo aspirare a rendere la pubblica amministrazione più efficiente anche nel Mezzogiorno d'Italia e

perché le politiche di *austerity* e il blocco delle assunzioni negli ultimi vent'anni le hanno desertificate e ci sono tanti piccoli Comuni che hanno difficoltà a partecipare a questa fase attuativa.

che stimolino l'aggregazione dei piccoli Comuni a partecipare insieme alla fase attuativa, altrimenti la partita rischia di essere difficile, soprattutto in alcuni territori e nelle aree interne. ormai la vocazione del legislatore, anche nella fase attuativa di strumenti finanziari, di immaginare che l'Italia sia solo città metropolitana; purtroppo non è così. L'Italia è il Paese dei piccoli Comuni e dobbiamo provare a tenere dentro a questo grande programma di innovazione del Paese tutte le piccole comunità, che devono contribuire; dev'essere un'operazione che ci consenta di rendere

Abbiamo davanti un appuntamento importante. Siamo riusciti, con una battaglia parlamentare, ad avere anche la garanzia che una quantità di risorse vadano al Sud. Qualcuno ha storto il naso rispetto a questo tema, ma credo che sia un elemento dirimente. D'altro canto, una delle questioni era quella delle differenze territoriali, oltre che a quelle di genere e generazionali. La parte che di questo provvedimento mi convince molto è quella che rafforza il ruolo del controllo parlamentare, che noi eserciteremo con ogni forma possibile e con ogni strumento, perché abbiamo la necessità di verificare in corso d'opera se gli obiettivi sui quali ci siamo impegnati vengono progressivamente raggiunti e se ci aprono una prospettiva. Concludo su questo: per me il PNRR è un cambio di approccio metodologico. Dobbiamo tornare a pensare con la prospettiva dell'intervento che programma i suoi risultati da qui ai prossimi vent'anni. Non dobbiamo più immaginare di utilizzare gli appuntamenti con la programmazione economica come quelli in cui calibriamo le risorse nell'ultimo miglio, con progetti spesso datati e nei cassetti dei Ministeri. È una sfida che abbiamo davanti e che dobbiamo affrontare tutti insieme. Sono però convinto che, come Parlamento, riusciremo a dare un ulteriore contributo, come abbiamo fatto qualificando il piano che poi Bruxelles ha

sono orgoglioso di intervenire oggi su un argomento così importante e quindi di fare il battesimo della mia presenza in Parlamento

abbia come obiettivo il bene del nostro Paese Italia. È una premessa che mi sento di fare perché il momento è così delicato che richiede una presa di coscienza comune, un'unità di intenti quanto mai necessaria e autorevolmente rappresentata rappresentata sempre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, specialmente in questi giorni, che ci vedono purtroppo molto molto preoccupati per la crescita dei contagi. Permettetemi di ringraziare il Governo per il fondo di 150 milioni di euro

che l'azione intrapresa, proprio con i fondi del PNRR, ridarà finalmente il ruolo che merita a un settore che, a mio avviso e come hanno ricordato i colleghi precedentemente, ha straordinarie potenzialità l'economia del nostro Paese. Ecco perché, onorevoli colleghi, è giusto ricordare che ci sono ancora situazioni problematiche, sulle quali non si è fatta, a mio avviso, necessaria riflessione. Queste incertezze rischiano, se non corrette in tempo, di pregiudicare quanto c'è di buono in questa manovra di bilancio, che dobbiamo approvare domani. Mi riferisco a una zavorra che pesa inesorabilmente sulle imprese italiane un limite alla loro crescita che è ben noto sia al Governo sia al nostro Parlamento. Parlo del peso delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti ai quali le imprese hanno avuto accesso prima della pandemia. Voglio ricordare che prima della pandemia, nel 2019, tantissime imprese italiane realizzarono con mezzi propri, soprattutto a mutui e finanziamenti, ingenti investimenti strutturali. Attenzione, colleghi, qui parliamo di imprese virtuose, che magari nei mesi più bui della pandemia, quando le attività produttive erano ferme e le saracinesche erano abbassate, durante il *lockdown*, hanno anticipato responsabilmente la cassa integrazione ai propri dipendenti per sopperire alle lentezze burocratiche. Cosa possiamo fare? Ecco, è necessario e urgente che il Governo - faccio qui un appello alla Sottosegretaria nel prossimo provvedimento economico intervenga a favore delle imprese affinché la moratoria delle rate dei mutui in conto capitale sia spostata al 30 giugno 2022.

Penso che tutti vogliamo che le nostre imprese continuino ad assumere e a produrre in Italia. Quello che vogliamo tutti è che l'Italia resti stabilmente nei Paesi con maggiore crescita, come adesso, lasciandosi quindi definitivamente alle spalle i tempi non troppo lontani in cui era fanalino di coda sulle riforme, sul PIL e sull'occupazione. Vogliamo un Paese prospero e forte e possiamo riuscirci nella misura in cui saremo in grado di spendere bene e nei tempi dovuti i circa 200 miliardi di euro europea, da qui al 2026, per il PNRR, un piano che - purtroppo - le Commissioni parlamentari del Senato non hanno avuto tempo e modo di approfondire per apportare miglioramenti.

i progetti, per poi vedersi attribuita la relativa responsabilità dei lavori, della loro esecuzione, dei collaudi e delle rendicontazioni delle spese per la concreta messa in opera. Da qui arriva la mia preoccupazione - che penso sia anche la vostra e di tanti italiani - sul fatto che gli enti locali

ma una riflessione fondata, dal momento che i fondi del PNRR rappresentano un *unicum* nella storia dell'Europa unita, come la pandemia che stiamo attraversando.

è che enti territoriali meno efficienti ed efficaci di altri, che sono concentrati soprattutto in alcune aree del Paese, ovvero al Sud, non siano in grado di spendere queste risorse. Sarebbe un dramma se il Piano nazionale di ripresa e resilienza, invece di unire il Paese, acuisse le distanze e il *gap* tra territori ricchi e territori poveri, fra aree sviluppate e aree arretrate. Sarebbe paradossale se se le parti dell'Italia che hanno maggior bisogno delle risorse del PNRR fossero, alla fine, quelle che riceveranno di meno, proprio per la scarsa capacità di gestione. Sarebbe paradossale se il Piano, che è nazionale, si rivelasse alla fine parziale e gli investimenti pubblici andassero solo a una parte del Paese. Tutti ci auguriamo che l'Italia possa ottenere e spendere, fino all'ultimo euro, questi 200 miliardi, ma non sarebbero soldi spesi bene, se alla fine ci trovassimo con un'Italia a due velocità. Per evitare questo scenario, è vitale il potenziamento delle infrastrutture al Sud. Su questo tema c'è una fortissima attesa da parte di milioni di cittadini e imprese e dev'esserci la massima attenzione da parte nostra. Al giorno d'oggi, i capitali si spostano con un *click*, ma le merci e le persone, inclusi i turisti, no. Ecco perché il Sud non può mancare quest'occasione per colmare il ritardo infrastrutturale. Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. L'auspicio è che, alla fine della realizzazione del PNRR, avremo un'Italia più moderna in tutto e - cosa ancor più importante - dappertutto e che si vada tutti insieme e alla stessa velocità verso un futuro più florido. Signor Presidente, ieri sera, libero dalle incombenze della legge di bilancio, essendo stato chiamato a esprimermi sul decreto di attuazione del PNRR (per gli amici e io ovviamente sono tra questi - il decreto *recovery*), ho aperto, con senso di responsabilità verso quest'Assemblea (per la quale provo la stessa riverenza che mi pervadeva quando, per la prima volta, vi entrai nel marzo 2018), il *dossier* elaborato con la consueta diligenza dagli Uffici studi parlamentari. L'ho aperto e subito richiuso. Non so se 483 pagine siano troppe o troppo poche per riassumere un provvedimento la cui elaborazione ha coinvolto ben 12 Ministri, si declina in 52 articoli e interviene con provvedimenti attesi e necessari, in ambiti che vanno dal turismo alle zone economiche speciali (ZES), all'istruzione universitaria, alla rigenerazione urbana, alle risorse idriche e al mercato dell'energia (ne tralascio altri, dato che mi sono stati assegnati dieci minuti a termini di Regolamento). Sicuramente queste pagine erano molte di più di quelle che un uomo del XXI secolo potesse assorbire nel risicato spazio che gli era concesso - che ci è stato concesso - per l'esame del provvedimento. Naturalmente, oltre che nel Governo, cui abbiamo dato fiducia, abbiamo totale fiducia anche nel lavoro che è stato fatto dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Diciamo così: fra due giorni scarteremo i regali sotto l'albero di Natale (spero di non urtare nessuna sensibilità, menzionando questa ricorrenza) oggi scartiamo in Aula questo pacchetto di provvedimenti, che giunge in qualche modo, anch'esso, come una sorpresa, nel senso che, con tutta la migliore buona volontà, essendo stati assorbiti dal disegno di legge di bilancio, pochi fra noi hanno potuto scrutare al suo interno. quindi di entrare nel merito, come hanno fatto con perizia e ammirevole spirito di sintesi i relatori e i colleghi che mi hanno preceduto. Mi limiterò a fare, a beneficio di chi ci ascolta, soprattutto da fuori, alcune considerazioni sul metodo, per stimolare, appunto, la discussione generale. Partirei da un dato: come le mezze stagioni, così sono ormai scomparse le doppie letture, soppiantate da eventi sempre più estremi. I decreti *omnibus* sono le bombe d'acqua che allagano le nostre Aule, mettendo a dura prova quella preziosa infrastruttura che è la Costituzione. Lo scollamento fra Costituzione formale e materiale è la prima cosa che mi ha colpito, quando sono entrato a far parte attiva e più o meno consapevole del processo legislativo. Il monocameralismo di fatto in cui operiamo mi ha portato, in un primo momento, a ricredermi sui giudizi politici, molto *tranchant*, che da profano avevo dato sulle proposte di riforma del collega Renzi; ho cominciato a pensare che il monocameralismo potesse non essere così male, se paragonato all'alternativa, così come la stiamo vivendo. Certo è, però, che l'esperienza di questo mese di dicembre mi ha portato a ricredermi ulteriormente. Alla domanda se una singola Camera avrebbe potuto sopportare peso di due provvedimenti ponderosi come la legge di bilancio e il decreto *recovery* la risposta temo sia no. *(Applausi)*. Il fatto è che la prassi di legiferare prevalentemente per decreti *omnibus*, una prassi verso cui si tendeva a vele spiegate già prima dell'emergenza, ma che l'emergenza ha consolidato, determina di fatto l'egemonia della 5a Commissione e la marginalizzazione delle altre Commissioni di merito, schiacciate su un ruolo puramente consultivo. In questo modo, però, fatta salva la facoltà di ogni collega di intervenire nei lavori di qualsiasi Commissione, si determina una sterilizzazione delle migliori competenze tematiche che questo Parlamento esprime, che non sempre riescono a essere coinvolte nell'esame di provvedimenti, cui potrebbero apportare un contributo significativo. La discussione in Aula, quindi, fatalmente assume la dimensione dello sfogatoio, in cui i colleghi delle Commissioni di merito, estromessi per cause di forza maggiore dall'analisi del provvedimento in Commissione, apportano un contributo che fatalmente si declina nelle forme del rammarico e della critica. Una soluzione va trovata, forse altrove, e trovarla è urgente. Non dobbiamo dimenticare che, per volontà sovrana degli elettori - che in modo, a mio avviso, paradossale si sono rivelati particolarmente ansiosi di ridurre i propri rappresentanti e quindi il proprio potere di rappresentanza, un po' come l'uomo che per castigare la propria consorte si sottopose alla stessa dolorosa operazione dell'Attis di Catullo *(Applausi)* - fra, al più, quindici mesi le Camere ripartiranno a ranghi ridotti e onestamente non so come potranno reggere l'eventuale protrarsi di una simile grandinata di decreti. C'è, poi, un altro problema di metodo, al tempo stesso più specifico, perché attiene alla materia europea, e più generale, che è quello di ricondurre a equilibrio, con onestà intellettuale, la narrazione sull'Europa. Lo scollamento fra Costituzione formale e materiale si combina in modo perverso con un altro scollamento, quello fra Europa narrata ed Europa reale, che, nella misura in cui genera aspettative eccessive, rischia di rivelarsi un *boomerang* per chi non lo contrasti, portando nel dibattito una voce di buon senso. Lo abbiamo già visto succedere con il meccanismo europeo di stabilità (MES). Ricorderete quando lo scorso anno questo fondo veniva acclamato come la soluzione decisiva, l'unica per finanziare il costo sanitario della pandemia; pareva che non ci fosse alternativa. Poi, invece, ne siamo venuti fuori - o, meglio, ne stiamo venendo fuori - senza attingere in modo improprio a un fondo nato per altre motivazioni. Aveva quindi ragione chi, come la Lega, esortava a non focalizzare tutto il dibattito e tutta l'attenzione su un unico strumento: problemi complessi non possono avere un'unica soluzione. *(Applausi)*. ma vale anche per la sanità, come i fatti stanno dimostrando. Cito il Partito Popolare Europeo, che quattro giorni fa su Twitter ci ricordava quanto qui, come Gruppo Lega, stiamo dicendo da aprile ed è consegnato agli atti di questo ramo del Parlamento, ossia che la vaccinazione non può essere l'unica risposta nella lotta al Covid-19, ma occorrono terapie. *(Applausi)*. Quindi, la notizia è che la Lega non è ancora entrata nel PPE, ma per fortuna il PPE è entrato nel buon senso della Lega. Ma, soprattutto, dove non c'è alternativa e non c'è politica, c'è la tecnica e dobbiamo interpellarci sulla tecnica, perché è quella stessa tecnica che ha consigliato per tanto, troppo tempo (e forse ancora oggi continua a consigliare, fra un canto di Natale stonato e l'altro), risposte semplici ma fallimentari, come l'austerità e altre più attinenti ai tempi che viviamo. Continuiamo a non ritenere molto opportuno presentare il *recovery* *plan* come l'unica soluzione, forse neanche come la soluzione decisiva alla crisi economica scaturita dalla pandemia. Si tratta naturalmente di uno strumento da sfruttare, visto che c'è, ma con piena consapevolezza non solo delle sue opportunità, ma anche dei suoi limiti; questa consapevolezza in Europa esiste. Continuiamo a essere perplessi sulla scelta fatta dal nostro Paese, con pochissimi altri e non fra i Paesi *leader*, di accedere allo strumento dei prestiti. La funzione dei prestiti è anticipare spese che non si hanno i mezzi finanziari per sostenere, ma in tutta evidenza - lo riconoscono anche i documenti della Unione europea, come le *in-depth analysis* sul Piano di ripresa e resilienza, pubblicate dalla Commissione le tempistiche ridotte del *recovery* mettono di fronte tutti i Paesi, non solo l'Italia, a un *trade-off* particolarmente insidioso, quello fra non assorbire tutte le risorse del *recovery* o farne un uso improprio, con sprechi e malversazioni, nel tentativo di spenderle comunque. Il decreto-legge all'esame incide con intelligenza su questi aspetti. Tuttavia vorrei qui valorizzare l'esigenza espressa dal collega Stefano di evolvere verso una visione programmatica di lungo periodo

Quindi, resta il punto che in questa fase il problema per il nostro Paese non è reperire mezzi finanziari, perché l'affidabilità internazionale di questo Governo ci tutela a sufficienza; il problema è spenderli e non è detto che la soluzione a questo problema possa arrivare per decreto-legge. Faccio un semplice esempio: ci sono voluti cinque mesi per trovare una *governance* alla principale stazione appaltante del Paese, l'ANAS, dopo l'infausto esordio di agosto che ricorderete. Questi sono problemi che oggettivamente incidono anche sulla capacità di spendere. Molto di quanto c'è da fare per sostenere la crescita del Paese, quindi, non dipende dagli altri e dalla loro supposta generosità, se tale è; dipende da noi, dalla nostra capacità di attivare finalmente un dialogo costruttivo e privo di pregiudizi tra la classe politica e la classe dirigente, che alcuni chiamano la classe tecnica del Paese. Un decreto-legge non può risolvere questo problema - che è culturale - ma può essere un'occasione per porlo, come ho fatto in questo intervento, sperando di non aver abusato del vostro tempo. *(Applausi)*. Signor Presidente, stiamo discutendo del PNRR e di come spendere queste risorse importanti. Ricordiamo il grande lavoro fatto dal precedente Governo e dal presidente Conte, che lottò per 90 ore consecutive per riuscire ad arrivare a questo risultato. Non possiamo dimenticarci quello che è stato. Anche con questo provvedimento, che stiamo analizzando,

perché a volte una delle due Camere non lavora perfettamente in sintonia con quello che dovrebbe essere lo spirito generale. In particolare voglio parlare dell'articolo 6, che tratta di alcuni tipi di opere pubbliche importanti, delle quali si è voluto modificare una legge approvata nel luglio scorso inserendo un comma aggiuntivo che, secondo l'intento, semplifica moltissimo il sistema. Ma noi dobbiamo anche preoccuparci che la semplificazione non vada a discapito della qualità. Quando si dice che possiamo mettere a gara lo studio di fattibilità tecnico-economica, che è il primo livello di progettazione, e su quello studio si lavora sulle Conferenze di servizi e si

Un'azienda di Stato può tranquillamente arrivare a fare un progetto definitivo, non credo sia così difficile; quindi si tratta solamente di lavorare con grande attenzione, bene ed efficacemente. Noi siamo convinti che le aziende di Stato di Stato lo possano fare tranquillamente, per cui ci chiediamo perché dobbiamo semplificare. Mi rendo conto che probabilmente parliamo della più grande infrastruttura ferroviaria da dobbiamo realizzare, ossia la Salerno-Reggio Calabria in Alta Velocità, ma siccome nel PNRR sono inseriti solamente i primi due pezzi, forse questo obiettivo si poteva raggiungere in altro modo. La cosa particolare è che questa disposizione, che esautora parzialmente la procedura della Conferenza dei servizi e i tempi della VIA, viene applicata anche a tutte le opere commissariate, nonché alle opere non oggetto di PNRR e del fondo complementare. allora: stiamo completamente stravolgendo il senso dei lavori pubblici, degli appalti, del modo di lavorare in questo Paese? In 8a Commissione stiamo

Naturalmente, lavoreremo in 8a Commissione per dare una delega al Governo che rimetta in piedi il sistema, in cui il progetto è garanzia per l'amministrazione pubblica e la sua esecuzione viene controllata dal direttore dei lavori, cercando di non eccedere nella sovrapposizione. quando i progetti vengono realizzati direttamente da imprese, associazioni tra imprese e professionisti e società di ingegneria, a volte l'interesse pubblico bisogna Il problema è proprio questo: quando vengono inseriti determinati passaggi alla Camera dei deputati e il Senato non ha la possibilità di correggere alcune misure che vengono inserite,

scrivere nel Regolamento del Senato che, ad eccezione dei casi di emergenza nazionale, il Governo non dovrebbe poter mettere la fiducia sui sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Forse sarebbe un po' forte, però, se vogliamo parlare di centralità del Parlamento, dovremmo iniziare a pensare a questo e dovremmo cominciare a togliere l'iniziativa al Governo per riprendercela noi. noi. Siamo assolutamente in grado di fare il nostro lavoro se lavoriamo per l'interesse collettivo, come sappiamo fare. A volte il Governo straborda un po'; forse dovremmo riprendere un po' la voglia di intervenire per evitare che succedano cose che poi non possiamo correggere. Ma le correggeremo nella

con una crescita fondata sulle tre direttrici fondamentali che attraversano tutto il PNRR, ma che sono anche nel disegno di legge di bilancio. Mi riferisco al sostegno all'innovazione tecnologica, alla transizione ambientale, spesso richiamata anche nel decreto-legge di attuazione del PNRR in termini di necessità di rispettare comunque e in ogni caso il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente

Ovviamente questo è uno degli assi portanti del PNRR, ma è rilevante anche per la legge di bilancio. Gli investimenti pubblici riguardano tutte le infrastrutture, materiali e immateriali,

che è fondamentalmente in larga parte spesa di investimento, e la legge di bilancio, che è in buona parte spesa corrente, si vede in modo molto rilevante proprio nei settori del *welfare* (scuola, sanità e istruzione). Vorrei ad esempio ricordare come al PNRR, che assegna risorse molto consistenti e assolutamente inedite per il nostro Paese ad un piano di costruzione e ristrutturazione degli asili nido, si affianchi nel disegno di legge di bilancio la scelta importante di finanziare con spesa corrente, che a regime arriverà circa al miliardo, il necessario il necessario finanziamento della parte corrente di spesa che rende possibile avere davvero gli asini, altrimenti avremmo solo scuole vuote e non avrebbe assolutamente senso. L'altro elemento di congiunzione fra i due interventi riguarda il sostegno agli investimenti privati,

cruciali per la realizzazione del piano, in particolare per quanto riguarda la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche per permettere a tutti di vivere la città. tuttavia importante, come è stato sottolineato, che ci siano - come ci sono, perché è previsto - piani differenziati, piani urbani integrati, che sono più appannaggio delle città più più grandi, le città metropolitane, ma anche l'attenzione, in un'ottica di equità e coesione territoriale, alla possibilità delle piccole comunità di partecipare attivamente a questo piano. Nel PNRR il ruolo del Parlamento è stato importante anche in questo campo, per sottolineare che, affinché questo sia possibile, è necessario continuare ad insistere, come si è già fatto più volte, con gli interventi che si sono succeduti. di permettere ai Comuni di contare su personale qualificato, non solo per la gestione e l'attuazione dei piani, ma proprio per la

riguarda la necessità di una massima trasparenza e di un monitoraggio valido e competente, con il rafforzamento del ruolo del Parlamento - come è stato detto - anche nell'ottica che ho già richiamato di una responsabilità collettiva.

l'equità intergenerazionale e l'equità territoriale. Per essere effettivamente conseguiti, tali obiettivi devono essere monitorati passo per passo.

a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

il PNRR è infatti quello strumento attraverso il quale il Parlamento, insieme al Governo,

senza rompersi e mi piace sottolineare proprio questo: assorbire gli urti senza rompersi. Abbiamo attraversato una crisi profondissima dalla quale, uniti, grazie al grande progetto portato avanti con l'Europa,

per costruire l'ossatura del Paese, un Paese ferito, ma non spezzato, che riesce, attraverso la resilienza, a ritrovare la forma adatta per essere pronto al cambiamento. il PNRR, un'offerta di importanti strumenti per raggiungere obiettivi di crescita e di sviluppo, dopo la drammatica esperienza della pandemia.

esce anche come modello di gestione di una pandemia mai vista prima, con regole mai viste, che l'Italia sembra aver creato e poi mutuato agli altri, tanto che altri Paesi stanno guardando al nostro. Noi, anche oggi, in un mondo e in un'Europa in grande difficoltà

desiderosi di tenere tutto chiuso, quando invece la grande forza nel marciare tutti insieme verso il raggiungimento di un obiettivo che portasse il Paese ad aperture graduali per non richiudere più, ha dimostrato di essere la strada giusta insieme alla grande campagna vaccinale. Tale campagna ha tenuto insieme anche la ripartenza economica del Paese. Siamo tra i primi al mondo per quanto riguarda il numero dei vaccini; siamo tra i primi ad essere riusciti a mettere in atto anche una sorta di regola che mantiene, nonostante i vaccini, il distanziamento, la mascherina e le misure di sicurezza e di protezione che non sono orpelli, ma strumenti fondamentali per poter garantire a tutti noi la ripartenza in sicurezza. Meglio si gestisce questa pandemia, minore sarà sempre l'impatto sull'economia nel caso di una nuova ondata. L'Italia è in questa buona posizione; abbiamo questa grande ripresa, la spinta dei consumi privati e degli investimenti. Proprio grazie all'attuazione inserite all'interno di questo decreto e di queste norme avremo strumenti capaci di farci fare un salto maggiore, di darci l'agilità necessaria affinché questo cambiamento di forma e questa resilienza siano complessivi. La crescita chiaramente è l'ingrediente essenziale e l'uscita dalla crisi deve andare di pari passo con queste politiche che aiutano ad aumentare la produttività e lo sviluppo economico. La crescita è anche la strategia migliore per per ridurre il male endemico del nostro Paese, che è il debito pubblico. Il percorso del Piano nazionale di ripresa e resilienza sta entrando proprio nella fase viva dell'operatività e dei fatti e sappiamo che questo piano complesso richiede anche una classe dirigente preparata a tutti i livelli sui territori. Ne abbiamo bisogno come il pane e stiamo vedendo in gli interventi che i nostri enti locali, Comuni e amministratori stanno facendo. Penso che il compito del Parlamento sia proprio quello di essere vicino a tutti gli amministratori locali, accogliendo le loro richieste, preoccupazioni e domande, aiutandoli a costruire le risposte giuste per essere sempre più efficaci nell'utilizzo di questi strumenti. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare contiene un grande pacchetto di misure necessarie ad affrontare anche le questioni più contingenti; ci sono aiuti per le imprese di diversi settori, dal turismo alla ristorazione, una serie di misure per accelerare la ripresa a ciò che può aiutare davvero l'Italia a trasformarsi in un Paese moderno a tutti gli effetti. Noi, come Partito Democratico, ci sentiamo in prima linea su questo. Sono molto contenta perché ieri in Commissione è stato approvato un ordine del giorno all'unanimità - lo abbiamo presentato noi, ma siamo contenti che sia diventato uno strumento di tutti - in cui abbiamo ribadito ciò che per noi è il punto prioritario di tutto questo lavoro.

con il Parlamento, che come abbiamo già visto non è supino al PNRR, ma vuole avere il suo protagonismo e lo sta rimarcando in tutte le fasi, questo confronto questo confronto sugli strumenti preposti alla valutazione d'impatto degli investimenti e delle riforme del PNRR. Si prevede, in particolare, un adeguato coinvolgimento della più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, sulla base delle migliori pratiche di valutazioni delle politiche pubbliche, al fine di vedere quali sono l'effettiva ricaduta e l'effettivo conseguimento degli obiettivi del Piano, a partire dai tre pilastri che in quest'Aula abbiamo ribadito più volte, ossia quelli che riducono i divari generazionali di genere e territoriali per garantire il più ampio coinvolgimento delle istituzioni territoriali. Noi ci siamo in quest'opera, insieme al Governo, perché siamo presenti sui territori e riteniamo

rispetto al quale vogliamo continuare a svolgere il nostro ruolo di parlamentari eletti dai territori, che riescono a portare

e quindi, a maggior ragione, bisogna mettere in campo tutti gli strumenti che ci permettono di assicurare una vera ripresa al Paese. Siamo stati i primi a discutere

Vorrei ricordare, a me stessa per prima, che i punti fondamentali del Next generation EU sono finalizzati ad avviare le transizioni più importanti, come la transizione ecologica, per rispondere non solo alle emergenze pandemica, economica e sociale, ma anche a quella climatica, attraverso uno strumento che ci faccia fare, tutti insieme, un salto in avanti. Ma il cuore del Next generation EU è la transizione ecologica intrecciata con la necessità di mettere in campo provvedimenti che rafforzino i territori e producano coesione sociale. Questi sono i due pilastri fondamentali,

di porre in essere anche prima dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia l'attenzione al reclutamento.

per poter realizzare e concretizzare i progetti. In questo decreto-legge vi è tutta una parte che riguarda il personale, che è molto interessante. Ovviamente sono tutte assunzioni a tempo determinato e io spero che per tempo ci renderemo conto che dobbiamo incrementare l'efficienza delle risorse

di tutte le opere si intervenga con la riduzione dei tempi per la valutazione all'impatto ambientale. Segnalo che anche la Conferenza dei servizi rischia di essere annullata, perché si procede con progetti non esecutivi ma di

il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere dannoso per l'ambiente. Allora, vorrei capire come misuriamo la sostenibilità di questi progetti; come misuriamo il fatto che debbano migliorare e non evidentemente creare danno; è evidente che restringere ulteriormente e pesantemente tutte le valutazioni per quanto riguarda l'impatto ambientale e la sostenibilità ambientale è rischioso. Quindi, mi auguro che su questo si ponga la massima attenzione, perché non possiamo assolutamente rischiare che

di vigilare e soprattutto di dare il proprio contributo. Speriamo che il rischio sempre più forte della marginalizzazione del Parlamento sia una parentesi che si chiuda in fretta. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole

Presidente, sottosegretario Guerra, onorevoli colleghi, è attraverso la buona riuscita dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che l'Italia potrà dimostrare se merita davvero i diversi elogi internazionali che arrivano in queste settimane, o se invece le grandi *performance* dell'ultimo anno sono state soltanto un episodio casuale e sporadico. Noi siamo convinti che l'Italia quelle lodi le meriti tutte: da un lato, perché adesso abbiamo una guida autorevole capace di dare credibilità al Paese, e poi perché siamo un grande popolo, composto da cittadine e cittadini, che, rispetto al dramma del Covid, ha saputo sacrificarsi molto di più che in altri Paesi e ha espresso un grande senso civico. Adesso è il momento di impegnarsi ulteriormente per dimostrare per primi a noi stessi dove possiamo ancora arrivare ed il PNRR è lo strumento giusto. Stiamo ricevendo ingenti risorse dall'Europa, quasi 200 miliardi di euro, ma non basterebbero tutti i soldi del mondo se quei soldi non venissero spesi bene, se non venissero allocati nei capitoli giusti, cosa che questo Piano meritoriamente sta cercando di fare. Come Italia Viva non possiamo che dirci soddisfatti per le previsioni di investimento in atto, a cominciare dalle risorse pensate a sostegno della parità di genere e della conciliazione tra mondo del lavoro e famiglia, con oltre 220.000 posti di asilo nido e 1.000 mense scolastiche; iniziative in linea con il nostro Family act, perché rappresentano una spinta al lavoro femminile, quel lavoro femminile che, se arrivasse ad eguagliare quello maschile, farebbe crescere il prodotto interno lordo del Paese, cioè la ricchezza nazionale, di ben 88 miliardi. Ecco che la *gender equality* non è solo un bel principio etico su cui disquisire nei convegni, ma anche una questione di crescita e di progresso generale. Del PNRR ci piacciono molto anche gli stanziamenti a favore delle infrastrutture: 25 miliardi in totale, con particolare attenzione al Meridione; soldi che rimettono in circolo lavoro, economia e mirano ad annullare i dislivelli territoriali, unendo l'Italia da Nord a Sud. Anche in questo caso si tratta di misure che sono in linea con quanto chiedevamo con il nostro Piano shock. Allo stesso modo, ci sentiamo in sintonia con il forte ambientalismo espresso dal Piano: penso agli stanziamenti contro il dissesto idrogeologico, voluti dalla ministra Bellanova già durante il suo precedente incarico al Dicastero per le politiche agricole e forestali, poi confermate dal suo attuale successore. Quante volte abbiamo lamentato la distruzione di splendidi paesaggi e borghi a causa di inondazioni, straripamenti, frane? Con le risorse messe a disposizione dal PNRR contrastiamo questa piaga dalle conseguenze spesso drammatiche. dunque strategici i quasi 80 miliardi che investiamo nella transizione ecologica, con interventi tanto ambiziosi quanto necessari: dalla riforestazione alla razionalizzazione della rete idrica e fognaria, dall'efficientamento energetico degli edifici al sostegno dell'economia circolare, dall'ultimazione del ciclo dei rifiuti all'aumento delle energie rinnovabili; tutte misure attraverso le quali la svolta ecologica diventa motore di sviluppo. modo, motore di sviluppo è destinato a diventare anche l'evoluzione digitale che, nel PNRR, occupa il 20 per cento delle risorse complessive. Investire in digitalizzazione ha un duplice effetto: da un lato, favorisce la crescita e, dall'altro, rende lo Stato più equo e più giusto, nella misura in cui diventa più accessibile. Non bisogna dimenticare che la mala burocrazia costa all'economia italiana oltre 60 miliardi all'anno: un costo che non possiamo più permetterci e che possiamo abbattere implementando il digitale. Modernizzare la pubblica amministrazione significa anche renderla più veloce e più connessa, cioè maggiormente al servizio dei cittadini. La necessità di digitalizzare non è un'opinione, non è un'idea visionaria, ma è un'urgenza più che attuale. Le risorse del PNRR che servono a innovare il Paese, signora Presidente, puntano di fatto ad annullare i *gap* ancora esistenti nella nostra società, cioè quegli squilibri che tuttora permangono e separano - ad esempio - le Regioni meridionali da quelle settentrionali o il mondo femminile dal mercato del lavoro. Noi vogliamo un'Italia in cui non ci debbano essere preclusioni *a priori*: non più uomo o donna, Nord o Sud; non più la scelta obbligata madre o lavoratrice, ambiente o sviluppo. Il Paese che vogliamo supera questi ritardi e lo fa proprio spendendo bene le risorse del PNRR. L'Italia del futuro vogliamo che sia inclusiva, verde, pulita, veloce. Allora virare verso politiche ambientaliste concrete piuttosto che verso l'utilizzo delle nuove tecnologie, allo scopo di semplificare, superare la burocrazia e snellire la pubblica amministrazione, non è più una scelta, ma diventa una necessità. Il PNRR, al contempo, è anche un gigantesco collettore di risorse, che purtroppo rischiano di fare gola ai malintenzionati e alle organizzazioni criminali. Ecco perché è opportuno che questo provvedimento preveda anche misure volte non solo a contrastare, ma anche a prevenire eventuali infiltrazioni mafiose, ad esempio attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo, che consiste nel fatto che il prefetto può adottare una interdittiva antimafia in via precauzionale laddove ritenga che siano sussistenti i presupposti. Le infiltrazioni criminali purtroppo sono un rischio più che reale e vanno attenzionate tanto quanto il rischio di non usare bene i soldi del PNRR. Se infatti permettessimo alle mafie di mettere le mani sul Piano, equivarrebbe ad aver sprecato questa grande occasione. Con il Next generation EU, l'Europa ha saputo reagire in modo straordinario al Covid, la più grave crisi dal dopoguerra ad oggi. Anziché arroccarsi su posizioni nazionaliste e fallimentari, l'UE è riuscita a mettere in campo misure fortemente europeiste inimmaginabili solo pochi mesi prima: la messa in comune del debito, la realizzazione di investimenti collegiali, la previsione di una sorta di grande Piano Marshall utile a far ripartire l'Unione tutta, così da far fronte all'emergenza sanitaria. L'Europa ha quindi capito il valore della solidarietà allo scopo di uscire dalla pandemia. Adesso sta a noi essere all'altezza della saggezza e della lungimiranza che l'Europa è riuscita a realizzare: o sapremo approfittare di questa *chance* alimentando con le risorse necessarie le riforme che stiamo mettendo in atto e che l'Italia aspetta da decenni, oppure torneremo a essere la cenerentola d'Europa. Non c'è una scappatoia e sarebbe una grave colpa se non riuscissimo a sfruttare bene l'occasione unica che la storia ci offre attraverso il *recovery plan* europeo. In conclusione, signora Presidente, il giudizio complessivo di Italia Viva sul PNRR non può che essere positivo, perché è in linea con le politiche portate avanti allora dal governo Renzi, così come con i valori fondanti del nostro programma: parità di genere, semplificazione, infrastrutture, ambiente, sviluppo. Sono interventi con i quali trasformiamo la crisi prodotta dal Covid in un'opportunità per creare crescita e progresso, superando i tanti nodi irrisolti, come burocrazia, scarsa produttività, dislivello tra Nord e Sud, territori disastrati, disuguaglianze di genere. Insomma, si tratta di un'opportunità che il Paese attendeva da tempo, anche perché consente di coinvolgere tutti gli attori della società civile (imprese, università, centri di ricerca, organi intermedi, terzo settore), mettendo in sinergia pubblico e privato. privato. Signora Presidente, se pensiamo a dove eravamo un anno fa, al piano presentato dal precedente Governo, alla situazione di stallo in cui eravamo sprofondati dal punto di vista sia economico che sanitario, e poi guardiamo all'oggi, ci rendiamo conto che quello scatto di reni all'inizio dell'anno, per il quale siamo stati tanto criticati, ma che ci ha consentito di innescare un cambio di Governo e di arrivare al voto odierno, oggi possiamo dire che è stata l'azione migliore che potessimo fare. Fare politica vuol dire trovarsi talvolta a un bivio, davanti al quale decidere se inseguire il consenso immediato o se agire per il bene del Paese per i prossimi decenni e segnare il corso delle cose. Noi abbiamo scelto il bene del Paese. Ci siamo fatti carico di scrivere una nuova pagina di storia. Questo PNRR ne è la prova e siamo certi che le risorse investite al meglio porteranno ancora più avanti l'Italia del futuro. *(Applausi)*.

il Gruppo Fratelli d'Italia non ha partecipato ai lavori delle Commissioni, né al dibattito in Aula sul decreto-legge relativo al PNRR per protestare contro il fatto che non ci è stato consentito un esame anche minimamente superficiale del testo arrivato in Senato. La nostra protesta riguarda sia i tempi che i modi con i quali il Senato è costretto a lavorare su provvedimenti che la maggioranza stessa definisce fondamentali. Noi non possiamo discutere, emendare o migliorare un testo che non conosciamo e non abbiamo potuto leggere. Il fatto, però, signor Presidente, che il Senato approvi un testo che non ha letto, che non ha compreso e non ha migliorato pare non interessi più a nessuno. Sicuramente non interessa a quest'Assemblea né ai capannelli che disturbano chi sta parlando,

Potevamo intervenire in questo dibattito orecchiando qualcosa, facendo riferimento ad articoli di stampa, copiando cose che hanno detto altri, oppure leggendo cose che altri scrivono senza magari comprenderle, ma credo che questa non sia la funzione cui siamo chiamati come senatori della Repubblica. Presidente, approfitto anche di questo intervento per segnalare il fatto che in Senato, all'approvazione di questo decreto-legge così importante, non è presente in questo momento alcun Ministro competente per la materia. Con tutto il rispetto per la sottosegretaria Guerra qui presente e per la ministra Stefani, a cui naturalmente va il nostro rispetto per il ruolo che interpreta come Ministro per le disabilità, ci aspettavamo un confronto almeno finto - signor Presidente, mi scusi - con qualche Ministro competente sul PNRR. Ma non c'è nessuno, e basta guardare i banchi del Governo. Questo è il dibattito del Senato sul piano fondamentale per il futuro del Paese:

Naturalmente tutto questo non disturba minimamente la coscienza e l'attività dei Gruppi di maggioranza, ma abbiamo il diritto di ricordarlo. Si è detto che l'accelerazione dei tempi deriva dal fatto che ci sono delle emergenze da rispettare, perché il PNRR deve entrare in vigore e ci sono degli obiettivi europei da raggiungere. Il ritardo con cui

Ricordo anche, soprattutto ai colleghi del Partito Democratico, che nel 2019 - quindi non un'era geologica fa ma due anni or sono - il Partito Democratico, a fronte del fatto che il Governo giallo-verde di allora aveva posto la aveva posto la fiducia sul maxiemendamento alla legge di stabilità, non solo protestò in maniera molto accesa, ma fece ricorso alla Corte costituzionale, per denunciare la violazione della libertà del Parlamento e del diritto-dovere del Parlamento di esaminare i testi della legge di stabilità. Dov'è finita quell'indignazione, colleghi del Partito Democratico? Adesso tutto va bene? Adesso va bene approvare il PNRR e porre la questione

a questa enfasi fa riscontro l'azzeramento del ruolo del Parlamento, che su questo Piano si dovrebbe esprimere, tentando di migliorarlo e perlomeno conoscendolo integralmente. Signor Presidente, il problema è che stiamo stiamo discutendo, come se fosse una sciocchezza, della trasformazione di questa Repubblica e del fatto che questa è una Repubblica parlamentare - come ci spiegano sempre i colleghi di maggioranza - soltanto quando si tratta di di difendere e giustificare i ribaltoni, i Governi multicolore e i cambi di maggioranza. *(Applausi)*. Allora è una Repubblica parlamentare! Quando invece si tratta di discutere di questioni importantissime, cessa di essere una Repubblica parlamentare e diventa di fatto una Repubblica presidenziale, semipresidenziale o come volete chiamarla. E lo dice uno che,

presidenziale e la trasformazione delle Costituzione senza che nessuno ne sappia nulla, nel silenzio generale o nel consenso generale di coloro che si stracciano le vesti, quando invece in Parlamento

con la differenza che quella che prima era una tendenza è diventata di fatto una deriva incontrollata e incontrollabile, che pare non interessare nessuno, nemmeno coloro che dovrebbero vigilare su tale deriva. Ricordo velocemente

individuali delle persone e le libertà costituzionali, senza nemmeno coinvolgere il Parlamento. C'è voluta una fortissima protesta, soprattutto di Fratelli d'Italia, per costringere il Governo perlomeno a portare, con decreti, nelle Aule del Senato e della Camera quei testi. Poi i decreti sono diventati piogge di decreti; poi i decreti a raffica; poi i decreti *matrioska*, e cioè un decreto che contiene un altro decreto, che contiene un altro decreto. E ancora: i decreti con la fiducia; e poi i decreti, con fiducia in prima lettura, che contengono centinaia e centinaia di articoli da approvare in poche settimane; poi i decreti con fiducia in prima lettura con centinaia di articoli *omnibus*, con dentro tutto e il contrario di tutto, dalle bollette del gas ai corsi di psicologia, salvo il fatto che il Parlamento su quello non poteva toccare palla. Tutti gli emendamenti, infatti, erano tutti considerati inammissibili

della tutela del Parlamento, sarà difficile ripiantarli, perché, una volta che la deriva vince e stravince, non c'è più spazio per nessuno. In conclusione, io vorrei dire soltanto che lo stato di emergenza in questo Paese è diventato stato di eccezione, con tutta la gravità che questo comporta. Faccio riferimento a quanto detto da un costituzionalista non certo di destra, Michele Ainis, che ha detto che, in questo momento, il generale Figliuolo vale più di mille parlamentari. parliamo del PNRR. Vorrei ricordare, a coloro che ci hanno accusato di essere euroscettici ed eurocritici, che il PNRR arriva dopo che noi, al Parlamento europeo, abbiamo condotto una battaglia contro il MES. Qualcuno si ricorda del MES? Ricorda che si diceva che gli ospedali avrebbero chiuso se non prendevamo i soldi del MES? MES? Ricorda gli appelli sulla gravità delle posizioni di coloro che non accettavano il dogmatismo europeo sul MES e sulla rigidità dei piani di *austerity* sul Patto di stabilità? *(Applausi)*. aver testimoniato una visione controcorrente e libera siamo noi. E questo dovrebbe insegnare qualcosa rispetto al fatto che in Parlamento serve una voce libera e controcorrente: serve al Parlamento e serve soprattutto al Paese, anche in una giornata triste come questa, signor Presidente, in cui, per la prima volta, nella storia della Repubblica, il Senato voterà due fiducie in dodici

colleghi, l'imponenza del provvedimento che andiamo a votare oggi, per il quale Forza Italia ha dato un contributo essenziale di collaborazione nei lavori della Camera, è testimoniata dalla notizia di pochi minuti fa, delle ore 11,30 circa, dalla quale risulta che è stata posta la firma, da parte del MEF e della Banca europea degli investimenti,

avremo 500 milioni che andranno a coprire tutte quelle partite del turismo che sono state già elencate nel corso della discussione generale. Non solo: abbiamo anche circa 278 milioni per la rigenerazione urbana,

che va ovviamente seguita con attenzione. Quali sono i pilastri fondamentali, che hanno visto - come vi dicevo - un lavoro parlamentare molto attento alla Camera e molto attivo da parte del mio Gruppo, che esprimeva uno dei relatori? Del turismo e della rigenerazione urbana ho detto. L'altro pilastro fondamentale è quello degli enti locali.

previsti 30 milioni per le assunzioni nei piccoli Comuni e una serie di assunzioni che riguardano le questioni relative ai supporti che deve avere la stessa struttura finanziaria ed economica del Ministero. Un altro pilastro - vado a volo d'angelo e cito dei punti essenziali - è la partita del digitale. All'interno di questo provvedimento c'è una parte importantissima che Forza Italia ha sostenuto convintamente ed è quella della conoscenza digitale in tutte le scuole.

un quarto pilastro che vorrei sottolineare e di cui non vi sfuggirà l'importanza. Anche su questo il lavoro parlamentare e del Gruppo è stato rilevante.

ci saranno le stesse modalità semplificate previste per il PNRR. Capite da soli ciò che significa in termini di accelerazione

mafiose; una serie di norme sempre introdotte da Forza Italia che modificano l'interdittiva antimafia; la parte

Sapete che sono state fatte delle procedure accelerate per venire incontro alle imprese che hanno problemi tramite le camere di commercio.

Abbiamo anche una norma che prevede che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio, debbano indicare le priorità per i processi penali.

rotta di collo per il riparto dei fondi. È stato fatto lo schema di decreto per le reti idriche (900 milioni distribuiti);

l'ultimo, di 450 milioni per i ponti e i viadotti. Vi ricordate i ponti e i viadotti dell'inizio della legislatura? Il riparto è stato fatto adesso, perché chiaramente c'erano le risorse.

in conferenza stampa è stato dato l'annuncio di uno dei bandi più importanti, quello che riguarda i borghi. Si tratta dunque di uno strumento importante

un testo che, introducendo semplificazioni delle procedure e lo snellimento della macchina amministrativa, dovrebbe essere un tassello fondamentale per la ripartenza dell'Italia dopo un 2020 e anche un 2021 che ci hanno visto e ancora ci vedono impegnati tutti nella crisi pandemica. una guerra che ha provocato tanti morti, che stiamo combattendo con armi diverse, certamente con i vaccini, ma soprattutto con i nostri sanitari, medici e infermieri, donne e uomini delle Forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, i sindaci e tutti coloro che si sono impegnati per superare questo periodo che ha portato il PIL dell'Italia nel 2020 ad un Gli ambiti di intervento toccati dal decreto sono tanti. Ne elenco qualcuno, a partire dal rilancio del settore turistico, ricettivo, fieristico e congressuale, prevedendo crediti d'imposta, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Agenzie di viaggio e *tour operator*, piscine, complessi termali, porti turistici, parchi acquatici, parchi tematici in generale e poi gli stabilimenti balneari sono destinatari di molte misure grazie all'azione del ministro Garavaglia *(Applausi)*, un super-pacchetto turismo con 2,4 miliardi stanziati per sostenere in modo importante un settore duramente colpito dalla pandemia. Vengono semplificate le procedure di approvazione del contratto di programma tra MIMS e RFI per ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari necessari per potenziare i collegamenti Nord-Sud e Est-Ovest nel nostro Paese. Viene previsto un piano di azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, per la ricognizione e riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale. Si introducono norme relative alle attribuzioni di contributi statali ai Comuni in materia di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, valorizzazione del territorio e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico. Si introduce, come chiesto a gran voce dalla Lega alla Camera dei deputati, il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Non è più accettabile infatti che oggi un'impresa debba fallire perché non incassa i crediti dallo Stato. Aspettiamo alla prova dei fatti l'efficacia di queste misure che dovrebbero mettere in grado il Paese e tutti i soggetti attuatori, Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende di Stato e imprese private di mettere a terra, entro il 2026, 235 miliardi che finanziano azioni e progetti in diversi settori. Stiamo insomma lavorando per concretizzare l'attuazione del PNRR, nato dopo la pandemia, uno tsunami che ha fiaccato il nostro Paese e l'intero pianeta. pianeta. Non posso in questa sede non toccare ancora il tema del caro energia, un altro tsunami che ci sta travolgendo e che rischia di vanificare gli sforzi del PNRR.

è stato per troppo tempo irresponsabilmente sottovalutato e lo è ancora oggi, soprattutto dalle istituzioni europee. Il caro energia non è ovviamente solo italiano, ma l'Italia soffre di più perché paga scelte discutibili e inefficienze mai risolte. Le cause di questa drammatica situazione italiana sono da ricercare nel nostro particolare *mix* energetico e nell'eccessiva dipendenza energetica dall'estero. Il nuovo intervento in manovra da 3,8 miliardi per contenere gli aumenti in bolletta per il primo trimestre 2022 è stato necessario, ma non è sufficiente, occorre fare molto di più. I beneficiari sono 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese, ma piccole, medie e grandi imprese, soprattutto le energivore, sono in estrema difficoltà. Per loro finora nulla o pochissimo è stato fatto. *(Applausi)*. Ci sono anche i Comuni in generale le pubbliche amministrazioni che non hanno magari fatto un contratto di fornitura a prezzo fisso, che hanno bollette raddoppiate se non triplicate. I prezzi del gas e dell'energia elettrica sono ormai fuori controllo. Oggi, 23 dicembre, l'energia elettrica è data a 414 euro a megawattora che fa innalzare la media giornaliera dei prezzi di dicembre a 303. Pensate che a dicembre 2020 eravamo a 54 euro a megawattora, un valore in linea con gli ultimi anni. Siamo ad un aumento del 765 Il gas è allo stratosferico livello di 180 euro a megawattora, a dicembre 2020 era a 16,5; la percentuale di aumento la lascio calcolare a voi, cari colleghi. Gas e luce continuano a salire e peraltro il generale inverno deve ancora arrivare e non illudetevi che a primavera del 2022 i prezzi possano scendere ai livelli della primavera di quest'anno. Purtroppo i *forwards* dicono che fino al 2023 i costi del gas rimarranno alti. Le cause di questo dramma: certamente la ripresa economica *post* Covid, che ha innalzato la domanda di gas, le strozzature sulle offerte di gas di fornitura, le speculazioni nel mercato del gas e soprattutto nel sistema ETS di pagamento della CO2. Vi sono poi temi di geopolitica relativi a tutte le tensioni in corso tra Occidente e Russia, principale fornitore di gas in Europa e in Italia che, invece di stemperare, l'Europa sta aggravando. aggravando. Tra le cause, vi sono le tante, troppe scelte sbagliate fatte in Europa e soprattutto in Italia, in nome di un ambientalismo integralista che, sull'onda del *Green Deal* e della decarbonizzazione, ha tagliato gli investimenti sul gas, che è invece strategico nel ruolo di accompagnamento alla transizione ecologica. *(Applausi)*. Ha invece investito troppi soldi - e lo sta facendo tuttora - sulle energie rinnovabili, che hanno un costo elevatissimo per la loro mancata produzione quando non ci sono sole e vento. Sono tante le conseguenze e i rischi che si stanno manifestando e mentre in Europa continuano a litigare su quali misure adottare, la Commissione UE irresponsabilmente cancella il raddoppio del TAP, che avrebbe consentito la diversificazione degli approvvigionamenti. Forse a Bruxelles sperano che il fenomeno del caro energia passi da solo e non si rendono conto che questa crisi è sempre meno congiunturale e sempre più strutturale. strutturale. In questi giorni, per carenza di energia elettrica proveniente dalla Francia, da cui dipendiamo, e per scarsa produzione delle rinnovabili, si sono riaccese le centrali a carbone di La Spezia e Monfalcone, che dovevamo dismettere. Per i costi insostenibili avremo un'accelerazione delle sospensioni di attività delle imprese e lavoratori costretti alla cassa integrazione. Vedrete che strage già a partire dai prossimi giorni. Lunedì nella fonderia di Torbole, nel bresciano, ci sarà una manifestazione di carattere nazionale, con centinaia di imprenditori in particolare del settore *hard to abate*, per lanciare un disperato allarme ed evidenziare la situazione drammatica che stanno vivendo. Stanno saltando anche i venditori di luce e gas e, per evitare il *default*, occorre che il Governo, a cui mi rivolgo in questo momento, consenta loro di fruire del fondo di garanzia Sace. Lo tsunami è arrivato e manca poco al collasso del sistema energetico, con possibili *blackout.* I rischi che venga frenata la ripartenza *post* pandemia e che parta l'inflazione sono altissimi. Urgono pertanto iniziative. L'Italia non può più aspettare l'Europa, divisa e - dunque - inerte. *(Applausi)*. Sulla reintroduzione del gas nella tassonomia, stanno ancora ritardando. Nell'immediato servirebbe un'azione diplomatica su Putin perché rilasci più gas russo e in Italia occorre subito una cabina di regia, come proposto da Salvini, per definire subito nuovi tagli nelle bollette e - poi - misure strutturali. Occorre introdurre finalmente sgravi fiscali alle industrie energivore e dobbiamo assolutamente riprendere a estrarre più gas. Occorre decarbonizzare anche con la cattura e lo stoccaggio della CO2, tecnologia che - invece - la sinistra e il MoVimento 5 Stelle, con la complicità del Partito Democratico, hanno affossato in legge di bilancio. Non bisogna perdere il treno dello sviluppo del nucleare di ultima generazione, che è pulito e sicuro.

Altro che rivoluzione verde, sarà un disastro. Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione

Poi è arrivata la pandemia, che ci ha mostrato quanto non si possa tagliare in questi settori e quanto l'Italia fosse indietro rispetto agli altri Paesi europei in digitalizzazione, ricerca e sviluppo. Bisognava, quindi, invertire la rotta e, per farlo, l'Europa ha messo a disposizione uno strumento che è rappresentato dai fondi del Next generation EU, quel grande piano di investimenti pubblici - il più grande dell'ultimo decennio che per la prima volta è alimentato da un debito comune e condiviso. Di questi investimenti, che ammontano a 750 miliardi di euro, l'Italia ha ottenuto quasi un terzo. All'Italia, infatti, sono andati ben 209 miliardi di euro e questo solo grazie all'impegno e alla dedizione del Governo Conte II e, in particolare, del presidente Conte. Per ottenere questi fondi, Presidente, questi 209 miliardi destinati all'Italia, abbiamo operato in assoluta solitudine, con un'opposizione che utilizzava la pandemia per accrescere il proprio consenso elettorale. Dei 209 miliardi, 80 sono a fondo perduto. Questi fondi vanno a finanziare quasi 150 nuovi progetti e 66 progetti in essere e rappresentano la base del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che incarna in pieno la visione di futuro del MoVimento 5 Stelle, che si basa su tre assi: la digitalizzazione, la transizione ecologica e l'inclusione e la coesione. Esso si sviluppa attraverso sei missioni. La prima missione punta alla digitalizzazione del Paese, che non vuol dire solo usare nuove tecnologie, ma riorganizzare i processi per migliorare i servizi per i cittadini. Significa modernizzare la pubblica amministrazione, semplificare i processi, sburocratizzare. La missione 2 del PNRR è destinata alla transizione ecologica, transizione ecologica, che di certo non vuol dire nucleare, come ha detto il senatore Arrigoni. Transizione ecologica vuol dire transizione energetica, che stiamo realizzando anche grazie a quelle misure visionarie ideate dal MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*. Penso al superbonus, alle comunità energetiche, alla tutela della risorsa idrica, che potremo realizzare riducendo il rischio legato al dissesto idrogeologico, anche grazie a strumenti come la cartografia geologica, che abbiamo finanziato nel disegno di legge di bilancio. L'abbiamo finanziata ancora una volta da soli, e lo abbiamo fatto in memoria del nostro compianto senatore Franco Ortolani. *(Applausi)*. La missione 3 del PNRR è dedicata alla mobilità sostenibile, per ridurre quel divario infrastrutturale che esiste tra il Nord e il Sud e il Sud del Paese, che viaggiano da decenni a due velocità e non solo in senso figurato. La missione 4 destina fondi all'istruzione e alla ricerca. Con questa missione, Presidente, andiamo a potenziare il diritto allo studio, affinché sia davvero un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. Abbiamo innalzato la *no tax area* per le tasse universitarie, da 13.000 euro nel 2017 a 23.500 euro, in modo che tutti i nostri giovani possano realizzare i propri talenti. Abbiamo aumentato il fondo tempo pieno a scuola e questo perché la scuola diventi davvero un luogo di riscatto sociale, soprattutto per tutti i giovani che vivono situazioni di disagio. Abbiamo rafforzato il Piano asili nido e servizi per l'infanzia. Oggi, la media italiana di asili nido è del 25 per cento, con il Nord-Est al 33 per cento e il Sud appena al 12 Andiamo ad incrementare le competenze STEM, quelle competenze in materie scientifiche che devono stimolare soprattutto le donne ad intraprendere una carriera scientifica. Andiamo a stanziare più fondi in ricerca e sviluppo: ancora una volta l'Italia è fanalino di coda in Europa con appena l'1,4 per cento del PIL investito in ricerca e sviluppo, che invece rappresentano il motore per la crescita economica di un Paese. Abbiamo più che raddoppiato le borse di dottorato di ricerca, portandole da 9.000 a 20.000. La missione 5 è dedicata all'inclusione e alla coesione. Andiamo a potenziare le politiche del lavoro che sostengano soprattutto i giovani e le donne. Facciamo partire quella fase 2 del reddito di cittadinanza che deve portare i percettori di reddito ad entrare finalmente nel mercato del lavoro. Anche il presidente Draghi ha detto spesso che non ci può essere crescita economica per l'Italia senza coesione sociale, coesione che va rafforzata soprattutto al Sud, perché se riparte il Sud riparte l'Italia. Infine, la missione 6 è quella dedicata alla salute. La pandemia ci ha mostrato con chiarezza cosa mancava al nostro Servizio sanitario nazionale: mancava un filtro al territorio, mancava personale, mancava la digitalizzazione del sistema ed è su questi pilastri che stiamo costruendo la sanità del futuro. Allora davvero, Presidente, spero che questo 2022 rappresenti l'anno delle grandi riforme, un po' come è stato come è stato il 1978, un anno in cui il Parlamento ha approvato delle leggi che hanno cambiato profondamente la società italiana: penso alla legge che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, alla legge Basaglia e alla legge che ha regolamentato l'aborto. Anche allora, dal fermento sociale nasceva la richiesta del Parlamento di ottenere più tutele e di valorizzare la libertà e i diritti dei cittadini. Il MoVimento 5 Stelle, ancora una volta, è stato cruciale in questo percorso di cambiamento, perché sa essere all'avanguardia su questi temi. *(Applausi)*. Per realizzare il PNRR però grande senso di responsabilità e di collettività, responsabilità che il Parlamento ha dimostrato in questi giorni, perché solo grazie a tale responsabilità approviamo queste riforme in tempo così ristretto, ma non si può continuare a mortificare la prerogativa del Parlamento. Il presidente Mattarella ci ha esortato spesso a diventare costruttori di bene: questo dobbiamo essere. Questo Governo e le nostre istituzioni adesso hanno il dovere di dimostrare ai cittadini e all'Europa che di queste risorse sapremo fare buon uso e onoreremo questo impegno.

È un Piano per il Paese? Peccato che il Paese da tempo non sappia nulla, poiché lo avete tenuto all'oscuro grazie a una informazione che è la voce del padrone.

non interessa governare per il popolo; vi interessa governare per le globalizzazioni finanziarie, per le multinazionali. Ecco perché insisto: Draghi è profondamente un uomo della cultura di Goldman Sachs. Draghi punta e arriverà al Quirinale, perché c'è un disegno globale e globalizzante che deve essere compiuto. Questo è l'obiettivo: disintegrare la vera economia italiana. Con il PNRR, voi intrappolerete l'Italia; altro che rilancio. Ho sentito affermare che ci sono tanti soldi da spendere, ma spendere i soldi non significa di per sé arricchire il Paese e l'economia italiana. Gran parte dei soldi saranno spesi in economie straniere, quindi andremo ad arricchire le economie degli altri; ci prestano i soldi per spendere a favore delle economie degli altri. Pensate all'ecosostenibilità o allo *switch* sull'elettrico: compreremo auto elettriche straniere e rovineremo il distretto della componentistica dei motori. Il PNRR è lo schema futuro di una globalizzazione che fregherà il *made in Italy*. Che dire della rivoluzione digitale? Voi state creando le condizioni per la sostituzione dei lavoratori con l'intelligenza artificiale, con la robotizzazione: è il ritorno alla schiavitù attraverso il debito. Del resto, quanto vi interessi dei lavoratori lo abbiamo visto: proteggete sempre le multinazionali (l'abbiamo visto anche con il *green pass*). A voi piacciono i nuovi padroni globali e i lavoratori debbono tornare a un feudalesimo moderno. Per questo Draghi è il garante del PNRR per quel mondo; per questo lo manderete a fare il governatore dell'Italia al Quirinale.

di legge n. 2448, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento,

del 16 novembre scorso, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2469 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», collegato alla manovra di finanza pubblica. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo

la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis,* del Regolamento e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2021, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 6 ottobre 2021, ha dichiarato collegato al completamento della manovra di bilancio 2022-2024, tra gli altri, un disegno di legge recante «Legge annuale della concorrenza 2021». Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2022-2024, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio); termine che comunque, in base alla prassi consolidata, riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di collegato del disegno di legge. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata NADEF del 2021. Inoltre, considerato che il provvedimento risulta composto di 32 articoli raccolti nei seguenti 9 capi (Capo I finalit;, Capo II rimozione di barriere all'entrata dei mercati, regimi concessori; Capo III servizi pubblici locali e trasporti; Capo IV concorrenza, energia e sostenibilità ambientale; Capo V concorrenza e tutela della salute; Capo VI concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica; Capo VII concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori; Capo VIII rafforzamento dei poteri in materia di attività *antitrust;* Capo IX nomine nelle autorità indipendenti), esso appare coerente rispetto ai parametri della omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono altresì conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. sensi dell'articolo 126-*bis,* comma 2-*bis,* del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 2469 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Ai sensi dell'articolo 129, comma 2 del Regolamento, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Passiamo dunque all'esame della seconda sezione del disegno di legge (articoli da 200 a 219). Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge.

Signor Presidente, vorrei denunciare per l'ennesima volta i colleghi del Gruppo Forza Italia, che continuano a fare i cosiddetti Non è possibile che, con una larga maggioranza, si continui a votare per i colleghi assenti, che non vengono a lavorare in quest'Aula, insieme a tutti noi.

non è ancora possibile procedere alle previste votazioni. Pertanto, in attesa di ricevere la documentazione necessaria

e nella seduta odierna ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le dichiara valide: nella Regione Abruzzo: Alberto Bagnai, Gianluca Castaldi, Luciano D'Alfonso, Gabriella Di Girolamo, Nazario Pagano; nella Regione Basilicata: Agnese Gallicchio, Arnaldo Lomuti, Salvatore Margiotta, Rocco Giuseppe Moles, Pasquale Pepe, Vito Rosario Petrocelli; nella Regione Calabria: Rosa Silvana Abate, Giuseppe Auddino, Fulvia Michela Caligiuri, Bianca Laura Granato, Ernesto Magorno, Clotilde Minasi, Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori; nella Regione Emilia Romagna: Enrico Aimi, Teresa Bellanova, Anna Maria Bernini, Paola Boldrini, Lucia Borgonzoni, Maurizio Campari, Marco Croatti, Vasco Errani, Gabriele Lanzi, Daniele Manca, Maria Laura Mantovani, Michela Montevecchi, Matteo Richetti e Armando Siri; nella Regione Friuli Venezia Giulia: Franco Dal Mas, Raffaella Fiormaria Marin, Stefano Patuanelli, Mario Pittoni e Tatiana Rojc; nella Regione Lazio: Bruno Astorre, Nicola Calandrini, Monica Cirinnà, Loredana De Petris, William De Vecchis, Emanuele Dessì, Elena Fattori, Maurizio Gasparri, Francesco Maria Giro, Elio Lannutti, Alessandra Maiorino, Marinella Pacifico, Annamaria Parente, Gianluca Perilli, Mariarosaria Rossi, Gianfranco Rufa, Matteo Salvini e Luigi Enrico Zanda; nella Regione Liguria: Sandro Maria Biasotti, Elena Botto, Francesco Bruzzone, Matteo Mantero e Vito Vattuone; nella Regione Lombardia: Alessandro Alfieri, Paolo Arrigoni, Luigi Augussori, Alberto Barachini, Simone Bossi, Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Giacomo Caliendo, Eugenio Alberto Comincini, Gianmarco Corbetta, Vito Claudio Crimi, Alan Ferrari, Adriano Galliani, Tony Chike Iwobi, Francesco Laforgia, Gianpietro Maffoni, Simona Flavia Malpezzi, Alfredo Messina, Franco Mirabelli, Antonio Misiani, Tommaso Nannicini, Simona Nunzia Nocerino, Gianluigi Paragone, Daniele Pesco, Simone Pillon, Daisy Pirovano, Roberto Rampi, Alessandra Riccardi, Massimiliano Romeo, Giancarlo Serafini e Danilo Toninelli; nella Regione Marche: Rossella Accoto, Andrea Cangini, Giuliano Pazzaglini, Sergio Romagnoli e Francesco Verducci; nella Regione Molise: Fabrizio Ortis; nella Regione Piemonte: Alberto Airola, Giorgio Maria Bergesio, Giovanbattista Fazzolari, Lucio Malan, Mauro Maria Marino, Carlo Martelli, Mariassunta Matrisciano, Enrico Montani, Cesare Pianasso, Roberta Pinotti, Elisa Pirro, Maria Rizzotti, Anna Rossomando e Giacomo Taricco; nella Regione Puglia: Michele Boccardi, Maurizio Buccarella, Alfonso Ciampolillo, Dario Damiani, Daniela Donno, Vincenzo Garruti, Roberto Marti, Assunta Carmela Messina, Cataldo Mininno, Gisella Naturale, Dario Stefano e Luigi Vitali; nella Regione Sardegna: Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, Elvira Lucia Evangelista, Emilio Floris, Ettore Antonio Licheri e Michelina Lunesu; nella Regione Sicilia: Cristiano Anastasi, Giulia Bongiorno, Antonella Campagna, Davide Faraone, Barbara Floridia, Gabriella Giammanco, Mario Michele Giarrusso, Pietro Grasso, Cinzia Leone, Urania Giulia Rosina Papatheu, Giovanna Petrenga, Vincenzo Santangelo, Renato Schifani, Valeria Carmela Maria Sudano e Fabrizio Trentacoste; nella Regione Toscana, Caterina Bini, Caterina Biti, Francesco Bonifazi, Laura Bottici, Gregorio De Falco, Gianluca Ferrara, Andrea Marcucci, Barbara Masini, Tiziana Nisini, Achille Totaro e Manuel Vescovi; nella Regione Trentino-Alto Adige: Dieter Steger; nella Regione Umbria: Luca Briziarelli, Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Stefano Lucidi, Fiammetta Modena ed Emma Pavanelli; nella Regione Veneto: Andrea Causin, Vincenzo D'Arienzo, Giovanni Endrizzi, Andrea Ferrazzi, Giuseppe Massimo Ferro, Gianni Pietro Girotto, Barbara Guidolin, Andrea Ostellari, Nadia Pizzol, Daniela Sbrollini, Adolfo Urso, Gianpaolo Vallardi, Orietta Vanin e Cristiano Zuliani. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate le elezioni. Finalmente siete senatori in senso pieno.

Vi ringrazio dell'attenzione e dei festeggiamenti che avete rivolto rispetto alle vostre convalide, di cui si sentiva assolutamente la necessità. Sulla base di notizie di bene informati, sospendo la seduta fino alle ore 21,30, con ragionevole probabilità che le cose vadano bene. *(La seduta, sospesa alle ore

alle ore 21,34)*. Vi comunico che, con una ragionevole probabilità di buon esito, la seduta riprenderà alle ore 22,30. La seduta è sospesa.

Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3*-ter* del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo della prima della prima sezione del disegno di legge n. 2448 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che include le modifiche approvate dalla Commissione in sede referente e sul quale, acquisita l'autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia. In conformità all'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 23.

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge presentato dal Governo. Ai sensi degli articoli 102-*bis* e 128, comma 6, del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente,

una nuova finestra"). Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.

con cui abbiamo condiviso tante battaglie e tantissimi progetti. Bartolomeo Pepe è stato un convinto ambientalista, da sempre impegnato nelle battaglie ecologiste contro la Terra dei fuochi e contro lo sversamento di rifiuti tossici nell'*hinterland* napoletano. Nel corso degli anni ha organizzato diverse manifestazioni a difesa dell'ambiente; tra le tante battaglie ricordo anche la richiesta della istituzione di un registro tumori nella Terra dei fuochi. promotore delle istanze ambientaliste che lo hanno portato ad ispezionare diversi siti di smaltimento di rifiuti in Campania. Siamo veramente sconvolti da quanto accaduto. Ci stringiamo forte intorno alla sua famiglia e ai suoi cari, esprimendo tutta la nostra vicinanza.

Mi unisco alle condoglianze, esprimo alla famiglia la vicinanza mia personale e di tutto il Senato e invito tutti i senatori ad osservare un minuto di silenzio.

oggi approviamo una manovra di prospettiva, figlia di una corretta analisi della situazione e utile per gettare le basi per una crescita sostenuta anche dopo il 2022. Ne abbiamo discusso più volte in questi mesi: la vera sfida è scongiurare che l'Italia torni alla crescita striminzita del passato, ma si collochi stabilmente nella media Europea, anche per garantire la piena sostenibilità del debito pubblico, ma non solo. La crisi energetica, le tensioni geopolitiche, la spinta inflazionistica e l'andamento della pandemia si stanno rivelando minacce molto concrete. quindi positivi quegli interventi che puntano a mettere in sicurezza la crescita economica, a cominciare da quelli a tutela del potere di acquisto per le famiglie, con le risorse contro il caro bollette e le nuove aliquote Irpef che hanno il merito di guardare sia alle fasce più deboli e ai redditi più bassi, ma anche al ceto medio. Così come molto importanti sono le misure che puntano alla promozione e alla tutela del lavoro, dalle decontribuzioni per le nuove assunzioni, alla norma sulle delocalizzazioni, dove i Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro hanno trovato un compromesso efficace per tutelare l'interesse nazionale, ma senza per questo intaccare la libertà di impresa. Due elementi meritano una menzione particolare: il primo è una novità forse unica, ossia che più di un miliardo, circa il 2,5 per cento delle risorse complessive, viene destinato ai giovani. In questo senso ho apprezzato molto l'invito del presidente Draghi, affinché ogni intervento sulle pensioni tenga sempre conto di chi un giorno dovrà andare in pensione. È giusto quindi tutelare e costruire scivoli per i lavori usuranti, ma per il resto bisogna sempre procedere per ripristinare quel patto tra generazioni, che soprattutto sul fronte pensionistico troppe volte è stato infranto, Il secondo elemento è l'istituzione di un fondo specifico per lo sviluppo della montagna, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche qui, forse per la prima volta, la montagna gode di un approccio strategico, perché solo così si possono affrontare tutti i nodi e le questioni, dalla salvaguardia ambientale alle particolarità del sistema produttivo, fino alla lotta allo spopolamento. Per ora è solo un inizio, perché le risorse stanziate sono insufficienti spero anche che con i prossimi provvedimenti si trovi una soluzione per lasciare ai nostri territori le risorse avanzanti dai ristori per la montagna. La verità è che le misure nazionali sono arrivate molto dopo rispetto a quelle provinciali e quindi queste risorse sono più che mai necessarie, per compensare lo sforzo degli enti locali. Sulle questioni che riguardano le autonomie speciali, la misura più importante, sostenuta anche da altri Gruppi, è quella che prevede, per gli anni 2022-2024 il ristoro nei bilanci provinciali in caso di perdita del gettito, per via della riduzione Irpef. In particolare, gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale dovranno essere stabiliti entro il 31 marzo 2022, in un apposito tavolo tecnico convocato al MEF, con la partecipazione dei rappresentanti territoriali. di una norma significativa, non solo nel merito, ma anche perché ribadisce e rinnova la natura pattizia del rapporto tra lo Stato e le autonomie speciali. Altrettanto importante è il nostro emendamento, con cui si estende il regime di tassazione separata anche alle due federazioni di associazioni sportive della provincia di Bolzano, VSS e USSA. In questo modo si riconoscono queste associazioni sportive come enti erogatori di servizi sportivi. Bene poi l'approvazione della nostra proposta per la costituzione di fondi interprofessionali per la formazione continua, non solo a livello nazionale, ma anche a livello territoriale. Si favorisce così un miglior coordinamento su scala locale delle iniziative di formazione, con una più ampia visione strategica rispetto alle trasformazioni dell'economia e del mercato del lavoro. Tra gli altri nostri emendamenti ci tengo poi a ricordare la proroga a tutto il 2022 dell'esenzione dell'imposta di bollo per i tirocini formativi e l'interpretazione autentica in materia di imposta di registro, nel caso di trasferimento di proprietà di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, da assegnare a cooperative e a singoli privati. Ringrazio il Governo e la Commissione, con cui c'è stato un proficuo confronto, così come c'è stato sugli altri temi a valenza generale, dove non abbiamo fatto mancare il nostro contributo, dalla rimodulazione dell'IRAP ai *bonus* edilizi. In particolare sul 110 per cento è stato giusto mitigare la trasformazione normativa, per non penalizzare famiglie e imprese che avevano già programmato gli interventi. Oggi siamo chiamati a chiudere bene la stagione del 110 per cento, una misura cioè con un approccio anticiclico, ma che non può e non deve trasformarsi in una misura strutturale, per i costi ingenti, per il rischio frodi e per l'aumento dei prezzi che è davvero troppo alto. Merita invece una dimensione strutturale la platea degli ecobonus tra il 50 e il 65 per cento, che per il tipo di interventi hanno rischi minori e garantiscono slancio agli investimenti e alla modernizzazione del Paese. Bene anche la proroga del canone unico patrimoniale, con la proroga dei versamenti al 31 marzo, ma credo che si sarebbe potuto fare qualcosa di più: gli ambulanti, gli esercizi commerciali e la gastronomia sono quelli che per primi risentono dell'andamento della pandemia. Per come si stanno mettendo le cose, spero che si intervenga nuovamente per una proroga almeno fino al 30 giugno. Signor Presidente, con questa legge di bilancio si conclude un anno in cui la nostra economia ha dimostrato una grande voglia di ricominciare; e lo ha fatto anche nei momenti in cui l'ondata pandemica tornava a colpire duramente. È un lavoro che, come sappiamo, non si conclude qui. C'è da far partire velocemente i progetti del PNRR; c'è la legge sulla concorrenza, che può dare un ulteriore impulso sul terreno della competitività e del dinamismo del nostro sistema produttivo; e c'è, naturalmente, la necessità di accompagnare tutte le imprese su cui pende la vitale questione della mancanza di liquidità. Tutte partite che si possono vincere a condizione che si vinca quella contro la pandemia. I dati di questi giorni sulla tenuta dei vaccini rispetto alle nuove varianti ci inducono a un cauto ottimismo. Forse non ne stiamo uscendo, come speravamo di poter dire qualche settimana fa, ma non ci devono essere dubbi sul fatto che la strada è quella della scienza e dei vaccini. Tutto il resto, quindi, dall'uso dei tamponi e delle mascherine all'aperto, ad eventuali nuove restrizioni, deve ruotare attorno a questo perno: terze dosi ed una seria riflessione sulla necessità del 2G anche per i luoghi di lavoro, se non addirittura di 1G, ossia delle terze dosi. Di questo si dovrà discutere nelle prossime settimane: viene discusso a livello europeo e io penso che possa essere la vera possibilità per debellare questo virus. Il 2022 sarà un anno molto importante. Esso richiede la stessa determinazione e la stessa unità di intenti. La legge di bilancio che approviamo oggi è un tassello di grande importanza: la strada è ancora lunga, ma è sicuramente quella giusta.

quando si vota e si discute di una legge di bilancio, ci sono molti modi di guardare al testo. C'è chi fa il bilancio dell'anno:

L'Italia è di nuovo protagonista in Europa: non più tardi di oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato un articolo importante con il presidente francese, Emmanuel Macron, sulle regole del futuro del Patto di stabilità. Più in generale, il nostro Paese è tornato protagonista. Un anno fa eravamo in crisi, un anno fa chiedevamo una svolta e la svolta c'è stata. Dall'altro lato c'è la possibilità di guardare ai provvedimenti di merito. Per noi lo ha fatto la collega Conzatti molto bene, ma ancora il collega Steger qualche istante fa ha detto cose che condividiamo. Tuttavia, signora Presidente, limito il mio intervento perché resti agli atti, per esprimere un garbato, ma civile dissenso sul metodo che questo Governo ha utilizzato per il disegno di legge di bilancio. Onorevoli colleghi, in quest'Aula poche persone come me possono essere considerate persone che non hanno fatto mancare in questo anno il consenso al Governo. Io penso che il Governo Draghi sia stato, sia e sarà una benedizione per l'Italia. Tuttavia, *amicus Plato, sed magis amica veritas*: non si fa una legge di bilancio così. Lo abbiamo detto negli anni del presidente Conte e lo diciamo oggi qua. Non è accettabile che la legge di bilancio diventi la legge di bilancio delle due notti: una notte in Commissione, una notte in Aula. Non è accettabile, ma non per le motivazioni contenute nelle norme. Noi condividiamo la stragrande maggioranza dell'impianto normativo della legge e voteremo con convinzione a favore della questione di fiducia. Non è però accettabile che il Parlamento sia costantemente costantemente - ignorato nell'azione di Governo. *(Applausi)*. È un punto che riguarda tutte e tutti. Io in questa Aula guardo in faccia chiunque quando dico che bisogna superare il bicameralismo. Io ho perso il mio incarico perché volevo superare il bicameralismo. Quest'ultimo però si supera con una riforma della Costituzione, non con uno strappo istituzionale e non si fanno così le leggi di bilancio. Se non lo dicessi non sarei serio con quella che è stata la mia posizione del passato, del presente e del futuro. Allora parliamoci chiaro: non so se sia il Governo dei migliori, per me è uno dei migliori governi. Questa legge di bilancio, come metodo, è una delle leggi peggiori per come è stata fatta. L'ho detto perché restasse agli atti e perché il signor Ministro dei rapporti con il Parlamento prenda atto di una critica pesante sul punto di metodo che abbiamo avanzato e lo dico anche perché dagli errori si possa imparare per il futuro. per il futuro. Ci sono infatti delle considerazioni che il Parlamento lascia al Governo e alla discussione istituzionale. Sono settimane che diciamo che sulla terza dose bisogna fare di più e meglio. Sulla prima e la seconda dose siamo stati i più bravi di Europa. Siamo stati i Siamo stati i campioni d'Europa della vaccinazione nelle prime due dosi, ma poi ci siamo fermati e mentre il Regno Unito passava, a tre mesi di distanza, al richiamo della seconda dose, mentre la Francia passava, a quattro mesi di distanza, al richiamo della seconda dose, noi abbiamo continuato, forse per difficoltà di natura organizzativa, a rinviare l'appuntamento con l'anticipazione del richiamo. Sono punti che poi paghiamo in termini di aumento di contagi. Concludo sul punto, dal momento che non faccio un intervento di merito avendo la collega Conzatti spiegato molto bene le ragioni dell'apprezzamento di Italia Viva al disegno di legge di bilancio nei contenuti; bisogna avere la forza e il coraggio di dire con verità che o ci si ascolta di più e meglio o si rischia di perdere quella straordinaria finestra di prosperità e di positività che quest'anno l'Italia ha vissuto. Signora Presidente, tra un mese il Parlamento in seduta comune eleggerà il Presidente della Repubblica. Onorevoli colleghi, lo elegge il Parlamento, non lo eleggono i sondaggi, non lo eleggono le redazioni delle riviste internazionali, non lo eleggono gli editorialisti. È l'atto supremo del Parlamento in seduta comune, perché elegge l'arbitro per i prossimi sette anni. Questo è il livello della dignità istituzionale e costituzionale del Parlamento. Ogni tentativo di far venire meno la centralità del Parlamento rispetto all'ambizione, all'altezza e alla grandezza delle proprie responsabilità è un atto che in qualche modo rende più debole e più fragile il nostro sistema istituzionale. Sono entusiasta allora del fatto che si sia cambiato Governo, sono entusiasta del fatto che il Governo abbia prodotto dei risultati, felice del fatto che l'economia vada meglio e orgoglioso del fatto di aver concorso a questo cambiamento. Con la stessa franchezza però, un anno dopo, mi ritrovo in una notte a dover dire in questa Aula che non si fanno così le leggi di bilancio. Voteremo la fiducia, signori del Governo, siate all'altezza della fiducia che il Parlamento vi dà. In questo passaggio della legge di bilancio questo tipo di altezza è mancato, mi spiace non dirlo di fronte al Ministro dell'economia che ho conosciuto come valente Ragioniere generale dello Stato quando avevo responsabilità di Governo. Se avessimo fatto noi quello che è stato fatto con questo disegno di legge di bilancio, l'opposizione non ci avrebbe fatto entrare in Aula. Noi oggi pensiamo di poter e dover dire che per dare una mano all'Italia occorre essere più attenti al rispetto delle istituzioni perché la forma in democrazia è sostanza. Signor Presidente, parto anch'io dalle considerazioni del senatore Renzi. Noi invece siamo all'opposizione e vi facciamo entrare in Aula perché crediamo nella centralità del Parlamento. Non condividiamo quello che state facendo, il metodo che avete utilizzato non solo per questa manovra, ma anche per tutti gli altri provvedimenti che l'hanno preceduta. Se qualcuno cade dall'albero oggi e si rende conto di quanti sono stati i ricorsi alla fiducia anche sulle leggi di bilancio, forse è stato da qualche altra parte

Avete tutti dalla vostra parte e state abusando del consenso che avete non tra la gente, ma tra i poteri forti e che oggi vi consente di trattare il Parlamento a schiaffoni. Vi diciamo questo perché la manovra

maggioranza del Parlamento e hanno un unico scopo, ossia non favorire qualche parlamentare, ma semplicemente migliorare una manovra nata male,

senza un sostegno concreto per le imprese? Avevamo chiesto che fosse sancito il principio del "più assumi, meno paghi", ma nulla.

Ci siamo battuti perché il vaccino - importantissimo, ma non unico strumento per combattere questa pandemia - fosse accompagnato da una serie di iniziative, come la ventilazione meccanica negli stabili

Abbiamo cercato di risolvere il problema relativo agli autistici e lavorato sul superbonus, eliminando quelli spruzzi di ideologia con cui era nata questa manovra. Penso all'ISEE sopra i 25.000 altre cose che nascevano da un retaggio culturale sbagliato e da una visione distorta della norma del superbonus, che era nata per far lavorare le imprese e non per favorire qualcuno rispetto ad altri. Abbiamo chiesto che fosse istituito un fondo per le conseguenze avverse del vaccino, ma ciò non è stato possibile perché oggi - non nascondiamocelo - molta gente non si vaccina per la paura e la confusione che voi, con i vostri messaggi, avete generato nell'opinione pubblica. Non posso credere che in Italia esista una percentuale

Abbiamo chiesto che le cartelle esattoriali non fossero solo rinviate, rinviate e rinviate. Abbiamo chiesto la ristrutturazione e la rateizzazione del debito, per dare modo alle imprese e alle persone non solo di pagare tra qualche mese, ma anche di riuscire rateizzare dopo la scadenza. la scadenza. Non siete stati in grado di fare tutto questo, perché la manovra parte condizionata fortemente dal fatto che ancora persiste, viene rifinanziato e addirittura potenziato il reddito di cittadinanza. Ecco, il reddito di cittadinanza per oltre 8 miliardi di euro condiziona pesantemente questa manovra e lo fa ideologicamente. Nessuno è contrario al sostegno delle persone che non ce la fanno, però avreste dovuto prendere tutta la grande esperienza dei Comuni, che da anni ormai distinguono coloro i quali hanno realmente bisogno del reddito di cittadinanza da coloro che potenzialmente potrebbero approfittarne.

con milioni di euro dati a persone che ne abusavano. È questa vostra ideologia che oggi frena lo sviluppo, frena le imprese, frena la possibilità di abbattere il cuneo fiscale: 8,8 miliardi di euro sarebbero stati un'ottima risorsa per abbattere il cuneo fiscale, sia per i lavoratori che per le imprese. Voi, invece, continuate a tirare dritto, a fare manovre che accontentino un po' tutti, ma con una logica del ribasso, mai al rialzo. in questo Paese esiste oggettivamente un'emergenza. Però quell'emergenza siete voi, siete un Governo che oggi non è in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e siete peggio di questa pandemia. Vi auguro, però, buon Natale. Uso queste parole, non «buone feste» o «serene feste», come ho sentito anche in questi corridoi, perché è da qui che bisogna lanciare segnali chiari, anche a chi ci ascolta, su quali su quali siano le radici della nostra millenaria civiltà cristiana. Non potremmo altrimenti poi pretendere che un'Europa lontana e sorda le possa capire, se non siamo in grado di capirle nemmeno noi. Tanti auguri e buon Natale a tutti. Signora Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, di legge di bilancio predispone il nostro Paese verso due nuove sfide: in primo luogo, consolidare e rendere strutturale una crescita economica più alta rispetto al passato, tenendo insieme e saldando in un unico tempo la crescita con la coesione sociale; luogo, le connessioni nei saldi di finanza pubblica del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della nuova programmazione europea determinano un nuovo volto dell'Europa, che lasci al passato la stagione dei tagli lineari, della riduzione della spesa pubblica, del binomio "nuove tasse-tagli alla spesa" e presenti al futuro il rilancio degli investimenti, nella sostenibilità ambientale, nella transizione ecologica, digitale e sociale. Ecco le ragioni per le quali a noi non interessa mettere bandierine sulle singole misure, poiché le radici del Partito Democratico naturalmente corrispondono a questa grande sfida; un progetto importante per il futuro del nostro Paese e per il futuro dell'Europa. Lavoro, equità, sviluppo economico ambientalmente sostenibile non sono in contrapposizione con la coesione sociale, con l'apertura di un nuovo discorso comunitario, con la lotta all'evasione fiscale, con la riduzione delle disuguaglianze. Sono temi centrali, direi fondamentali, nel rapporto tra il centro e la periferia; sono al centro dell'agenda politica del Governo e del nostro Paese. al nostro esame, colleghi senatori, serve innanzitutto all'Italia per ripartire. Per ripartire abbiamo restituito centralità e importanza alla pubblica amministrazione, alle necessarie connessioni tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, elementi decisivi anche a legislazione invariata per dare piena attuazione alla sfida dell'Europa e al pieno utilizzo delle risorse. Il senatore Renzi ha posto un tema cruciale per restituire centralità al Parlamento: la nostra naturale funzione legislativa e di indirizzo ha teso negli ultimi decenni a smarrirsi di fronte ad un utilizzo eccessivo della decretazione d'urgenza. Però, diciamolo con chiarezza colleghi, mai come all'interno di una pandemia l'uso della decretazione si è rivelato indispensabile per attraversare e superare la crisi pandemica. durante la discussione sul disegno di legge di bilancio, diversi provvedimenti economici di altrettanta importanza strategica: mi riferisco al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle riforme necessarie per accompagnare il Paese fuori dalla pandemia e per consentire all'Italia di ripartire. Ovviamente il tema c'è, esiste e dobbiamo cercare nuovi metodi di lavoro. Dobbiamo capire che ci sono esigenze anche legislative da correggere: i tempi del disegno di legge di bilancio risentono inevitabilmente del passaggio della dimensione europea della nostra legge di bilancio. Il documento preliminare di bilancio viene presentato all'Europa con tempi probabilmente incompatibili con una doppia lettura. Dobbiamo lavorare a legislazione vigente nella correzione delle norme se vogliamo effettivamente restituire quel ruolo centrale al Parlamento, una volta usciti dalla crisi pandemica, nella riduzione anche della decretazione d'urgenza, che non può essere eccessiva, ma deve ricollocare il nostro Paese dentro il binario legislativo corretto. Ecco perché, lo diciamo con chiarezza, c'è fiducia nell'Italia, nonostante la crisi pandemica non sia alle nostre spalle, e i dati anche di oggi ci mostrano un'emergenza ancora presente e un impegno ancora necessario per superare questa crisi pandemica. C'è fiducia nell'Italia, tra le famiglie e le imprese italiane. C'è fiducia nell'Italia in Europa, perché cresce la propensione ad investire e la ripresa degli investimenti pubblici e privati rappresenta una strada importantissima per consolidare la crescita economica. Ma soprattutto, signora Presidente, abbandoniamo la presunzione dei due tempi: di un primo tempo necessario per costruire crescita e produrre ricchezza e di un secondo tempo per redistribuire la ricchezza prodotta per la coesione sociale e per contrastare povertà e solitudine. Se sapremo rilanciare gli investimenti e utilizzare al meglio i 320 miliardi tra PNRR e programmazione europea, restituendo centralità ed efficienza alla pubblica amministrazione, potremo finalmente progettare una crescita inclusiva, che non lasci sole le persone, i lavoratori, i giovani e le famiglie, ma che prevenga la solitudine, rispondendo in modo efficace alla povertà. Non conosciamo una strada alternativa alle riforme, se le riforme incontreranno nuovamente la dimensione popolare, cioè il consenso dei cittadini e non saranno rappresentate da artifici interni, lontani dalla dimensione popolare. Ecco perché è un disegno di legge di bilancio che non chiede ma dà, non chiede ma dà, che destina oltre 8 miliardi alla riduzione delle tasse. Ci troviamo a nostro agio all'interno di questa strategia, perché anche la riforma dell'Irpef ha salvaguardato la progressività, ha evitato l'appiattimento e le disuguaglianze e, soprattutto, ha mantenuto i principi fondamentali che caratterizzano il nostro sistema fiscale. La progressività non è una questione banale, non è un'ingegneria tecnica, ma è un elemento di equità e di giustizia per salvaguardare il principio di chi più guadagna, più partecipa ai costi per garantire la salute pubblica e l'istruzione pubblica. *(Applausi)*. Era giunto il momento di fare una scelta importante nella riforma dell'Irpef sul ceto medio. Non vogliamo evitare questa riflessione, dopo aver introdotto il reddito di cittadinanza, dopo aver lavorato per introdurre nel reddito di cittadinanza misure che noi riteniamo ulteriormente da correggere, perché la povertà abita nella dimensione territoriale e non si risolve con una carta di credito, perché la povertà richiede un lavoro dell'associazionismo, del volontariato, degli enti locali e non ci arrendiamo all'idea che non servano modifiche. Tuttavia, le risorse destinate al reddito di cittadinanza fino a pochi anni fa non avevano capitoli di bilancio sufficienti per affrontare il tema della povertà. Ecco perché era giusto intervenire in modo prevalente sul ceto medio. Ecco perché è indispensabile ricostruire la dimensione del ceto medio, favorendo i consumi interni, evitando di spingere verso forme di nuova povertà il il baricentro del nostro Paese, la capacità cioè di produrre ricchezza e di trasferirla nei consumi interni e nella crescita del nostro Paese. È stato importante salvaguardare il cuneo fiscale e investire sulla riduzione del costo del lavoro, come è stato importante eliminare l'IRAP in modo particolare per le tantissime partite IVA, per la piccola impresa, per il lavoro autonomo: una richiesta straordinaria che portiamo finalmente nelle condizioni di rappresentare un architrave importante della nostra economia. Ecco perché questa fiducia non va sprecata. Il Paese ci chiede stabilità, rigore, responsabilità. Dobbiamo continuare a lavorare per portare l'Italia fuori dalla dinamica pandemica e, soprattutto, dobbiamo consentire a questo Paese di non perdere la sfida dell'appuntamento con gli investimenti europei, con la transizione digitale, ambientale ed economica che - lo diciamo subito - ha bisogno di un piano regolatore dello sviluppo economico di questo Paese. Attenzione, colleghi, la transizione può anche spingere migliaia e migliaia di lavoratori verso forme di solitudine, migliaia e migliaia di imprese verso un futuro che può essere più complesso del passato. Ecco perché - lo dico con orgoglio - abbiamo ritenuto importantissimo lavorare, insieme a tutta la maggioranza, per rimettere al centro il tema del sapere, della scuola, dell'istruzione, delle politiche attive, della formazione. Non ci sarà un futuro per questo Paese se non rappresenteremo e non riprenderemo in mano il terreno della formazione, della scuola, di una scuola di qualità per tutti, di percorsi di formazione necessari per accompagnare la transizione. Diversamente, la transizione, anche quella digitale, ambientale e sociale, potrebbe spaventare e reintrodurre in questo Paese possibili conflitti se non riusciremo a definire bene le articolazioni del nuovo sviluppo industriale, di un nuovo piano di sviluppo industriale del nostro Paese. del nostro Paese. Dovremo riposizionare bene l'investimento nei saperi, nelle competenze, uscendo da una forma che troppo spesso anche sugli ammortizzatori sociali è di tipo assistenziale e non di tipo promozionale, attivo, formativo. Ecco l'importanza della riforma degli ammortizzatori sociali e l'importanza di questa legge di bilancio che non lascia soli i lavoratori; ecco perché abbiamo ritenuto importante rimettere al centro il lavoro come elemento fondamentale per costruire un futuro a questo Paese e per programmarlo questo futuro. Nella legge di bilancio ci sono questi elementi importanti. Come ho detto prima - e concludo, signor Presidente - questi elementi sono fondamentali, per noi naturali, nel sostegno al Governo, nella responsabilità di guardare al nostro Paese nell'interesse generale e, soprattutto, di investire in forme nuove affinché i giovani tornino ad avere fiducia nelle istituzioni, abbiano un accesso al lavoro che premi le loro competenze e non le sfrutti e le usi senza garantire contratti di lavoro importanti, regolari...

dopo una discussione che è stata certamente faticosa, ma anche molto ricca e ha dato anche molti contributi nel passaggio parlamentare. Non voglio sfuggire alle questioni che sono state poste poc'anzi, che hanno che hanno messo l'accento - penso all'intervento del senatore Renzi - sulla marginalizzazione, nei fatti, del Parlamento;

sono anche necessarie. Dico in premessa che abbiamo presentato emendamenti e riteniamo che quella norma sia certamente un passo in avanti, perché prima non avevamo assolutamente nulla, ma credo che sul lavoro c'erano anche la sensibilità e la possibilità di mettere in campo misure di cui si è discusso per molto tempo anche in questi anni, di fronte a un fenomeno che per l'Italia è stato ed è pericoloso e complesso come quello

per rispondere ai tanti lavoratori che in questo momento stanno ancora lottando e cercando di avere una possibilità di futuro. che non è soltanto e unicamente una questione di rivendicazione di poteri, ma vi è la necessità assoluta, per un Paese che vive e sta vivendo ancora un momento di difficoltà, di riuscire a mettere in campo tutte le risorse, le possibilità d'incontro e le discussioni

certamente è arrivata molto in ritardo all'esame del Senato - che ha degli elementi espansivi. Si colloca certamente in una fase positiva perché abbiamo dei segnali molto importanti (pensiamo alla crescita ma sappiamo anche che è un momento di passaggio, perché siamo in una fase ancora delicata. Purtroppo abbiamo una ripresa della pandemia, non possiamo ignorarlo,

le necessità che sono oggi di fronte a noi. Non siamo fuori. Non dobbiamo sederci, perché non siamo assolutamente fuori dal momento critico. Contemporaneamente questa manovra di bilancio presenta molti elementi e vorrei dirlo e vorrei dirlo a dimostrazione del fatto che il lavoro parlamentare è fondamentale, perché noi non stiamo qui soltanto per schiacciare i bottoni, ma per fare proposte, per articolarle, per mettere in campo le esperienze e il lavoro anche dei territori e di tutti

tutta l'Europa da una situazione difficile, affrontando la crisi pandemica e dando risposta anche all'altra grande crisi e all'altra grande emergenza di cui spesso ci riempiamo la bocca, salvo

perché la pandemia ha lasciato molti problemi. Contemporaneamente la dobbiamo affrontare facendo un grande lavoro per la trasformazione del Paese. Non bastano solo le riforme che annunciamo, ma abbiamo la necessità di pensare questo futuro e di costruirlo.

che sono trent'anni che non fa più politiche industriali e che non ha più un'idea di politiche industriali. Quindi spingere sulla transizione ecologica significa avere la capacità di mettere in campo, di dare le linee, di costruire, di dare incentivi e contemporaneamente di farsi carico di quelli che potrebbero essere i costi, da questo punto di vista. Con la manovra al nostro esame lavoriamo molto bene sulla scuola,

mettere in campo tutti gli elementi di coesione sociale che il Paese merita. Il nostro è un grande Paese, ha grandi potenzialità e su questo dobbiamo costruire insieme il progetto per il futuro.

Governo, come un anno fa ci ritroviamo in quest'Aula ad approvare una legge di bilancio in piena ondata pandemica, che in questi giorni e in queste settimane tiene sotto pressione il nostro sistema sanitario ed economico. Rispetto allo scorso anno c'è però una differenza sostanziale molto importante: questa volta abbiamo alzato un muro di difesa, che ci sta proteggendo dalle conseguenze più gravi di questa ondata, di questa nuova variante questo anno e in questa occasione abbiamo l'80 per cento degli italiani immunizzato con la doppia dose. È grazie a questo grande senso di responsabilità

che oggi riusciamo ad affrontare con relativa tranquillità questa nuova variante. La nostra campagna vaccinale è riconosciuta oggi come modello a livello europeo e a livello mondiale. La vita umana e l'economia si salvano con la vaccinazione di massa: dobbiamo ricordarlo sempre. Noi di Forza Italia non abbiamo assolutamente tentennato, non abbiamo mai avuto alcun dubbio, fin dal primo momento, sostenendo questi provvedimenti, che perseguono l'obiettivo principale, l'obiettivo più nobile, che è quello della salute pubblica degli italiani. È dall'insediamento di questo Governo, dopo la nomina del generale Figliuolo, che è avvenuto quel cambio di passo rispetto a una campagna vaccinale che stentava a partire. Gli italiani hanno compreso che senza solidarietà e senza un percorso comune non c'era la possibilità di contrastare il virus.

Quindi, continua il salto dell'economia verso i livelli precedenti all'emergenza economica. I dati del PIL li conosciamo tutti: con una crescita di oltre il 6 per cento, siamo in una fase espansiva. Questa fase espansiva si ripercuote in maniera positiva anche sui dati occupazionali. Se, infatti, vediamo i dati dell'ultimo trimestre, abbiamo finalmente un più 0,4 per cento. È chiaro che le previsioni economiche positive per il 2022 poggiano sul perdurare di una situazione di crescita, ma anche su una situazione, che noi abbiamo che noi abbiamo già creato in questo anno, di assenza di nuove restrizioni. Non possiamo più chiudere il Paese, non ce lo possiamo permettere. Di conseguenza, in questo momento particolare

Quindi, serve una cornice importante di sicurezza sanitaria, per avere appunto una strategia economica di ripartenza molto solida. Lo ribadisco ancora una volta, come ho già fatto in altri interventi in passato: fin dall'inizio, Forza Italia ha lavorato per coniugare e garantire al Paese sicurezza sanitaria, tutela del lavoro e ristori adeguati. a chiedere, qualche tempo fa, 100 miliardi di scostamento di bilancio per aiutare il nostro Paese: e avevamo ragione, perché poi di scostamenti di bilancio e di aiuti ne abbiamo dati ancora di più. Rivendichiamo, quindi, la nostra coerenza nella richiesta di provvedimenti che andavano e che vanno nella direzione delle famiglie e delle imprese che sono state travolte da questa emergenza. Lo facciamo attraverso misure che vedono il taglio e il rinvio delle tasse ed aiuti concreti. Da dieci mesi a questa parte, con il Governo in carica, il nostro contributo è diventato fattivo, decisivo. In tante norme di questa legge di bilancio c'è il marchio di fabbrica di Forza Italia impresso

l'Irap: abbiamo chiesto 10 miliardi, ne abbiamo ottenuti otto, ma oggi 850.000 aziende, imprese e persone fisiche, che hanno un reddito autonomo, non pagheranno più l'Irap. È un inizio e siamo impegnati a fare ancora di più nei prossimi mesi. *(Applausi)*. Il ceto medio era stato eliminato dai *bonus* e dagli aiuti. Non abbiamo fatto tanto: invece, con il taglio delle aliquote oggi aiutiamo, finalmente, il ceto medio a recuperare quel potere di acquisto che ha perso in tutti questi anni.

del pagamento delle cartelle era doveroso, a costo zero per lo Stato, ma lo dovevamo fare per gli italiani. È stata questa per noi una richiesta dirimente, che abbiamo vinto e ottenuto. La sicurezza, le Forze di polizia, gli stanziamenti e le risorse, le assunzioni e la tutela legale; anche questa è stata una battaglia di queste settimane e anche su questa abbiamo avuto ragione. I *bonus* edilizi hanno dato tanto alla nostra economia, bisognava continuare su di essi; 4,4 miliardi nei prossimi anni in aiuto agli italiani e soprattutto sulla casa, un investimento particolare dei nostri italiani. Per quanto riguarda le bollette elettriche e il gas, anche in questo caso avevamo chiesto un fondo di garanzia per aiutare gli italiani e le imprese, lo abbiamo ottenuto e realizzato,

abbiamo veramente lavorato tanto, siamo anche molto stanchi e affrontiamo l'ennesima nottata dopo le sedute notturne della Commissione bilancio. È stato un anno particolare, difficile e molto complesso, ma il percorso del Governo, declinato nel segno dell'unità, dello spirito di coesione e del perseguimento dell'interesse comune nella lotta al virus, più volte auspicato e indicato, con grande intuizione politica, dal nostro presidente Silvio Berlusconi *(Applausi)*, ha consentito di raggiungere i risultati messi oggi nero su bianco in una legge di bilancio che, come sappiamo, è l'atto politico fondamentale a cui riteniamo di aver dato un grande contributo con lo spirito di servizio, indossando tutti quanti noi, la maglia azzurra. *(Applausi)*.

il giudizio della Lega rispetto alla legge di bilancio è sostanzialmente positivo. Dispiace che i tempi siano stati troppo compressi a causa di un'approvazione tardiva della manovra da parte del Consiglio dei ministri e della concomitanza con la discussione alla Camera dei Deputati è stata quindi la difficoltà di analizzare gli emendamenti e le proposte avanzati da parte dei vari Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione. però nei contenuti di questa legge di bilancio. Il motivo principale è legato alla scelta e alla possibilità di ridurre la pressione fiscale; 8 miliardi di riduzione per noi rappresentano un segnale importante e finalmente, per la prima volta, l'Europa ha permesso al nostro Paese di utilizzare *deficit* per abbassare le tasse. È un precedente, una conquista di questo Governo, sicuramente grazie all'autorevolezza di Mario Draghi. Ricordiamoci che il *deficit* che siamo stati costretti a utilizzare nell'anno passato era riferito quasi esclusivamente a ristori, a manovre di sostegno e quindi non alla riduzione della pressione fiscale, ma ad inseguire i danni creati alla nostra economia dalla recrudescenza della pandemia.

Devo dire anche che, nella scelta di come ridurre la pressione fiscale, la Lega è stata protagonista nella trattativa all'interno della maggioranza. Siamo molto soddisfatti *(Applausi)* delle scelte che sono state fatte perché rispecchiano rispecchiano interamente il programma della Lega, le sue convinzioni e le sue valutazioni. Assistiamo ad una riduzione dell'Irpef per lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti. Assistiamo soprattutto all'abolizione dell'IRAP per i lavoratori autonomi, per le ditte individuali e le imprese familiari. Questa era l'impostazione in cui abbiamo creduto e che alla fine

il tentativo di arginare gli effetti negativi del caro bollette e del caro energia. Il Governo ha già stanziato, nella fase finale di quest'anno, importanti risorse quasi 4 miliardi di euro - per la riduzione di questi aumenti e investirà anche in questa legge di bilancio per l'anno prossimo. Questa è la nostra più grande preoccupazione,

in un certo numero di anni e che non si possano interrompere a metà percorso. *(Applausi)*. Gli emendamenti approvati vanno dunque proprio in questa direzione. Non si può lasciare il cittadino nella continua incertezza di norme approvate e successivamente modificate o abrogate. Questo è uno dei gravi problemi dell'attività parlamentare italiana, che non dà certezze ai cittadini. Con l'azione emendativa svolta in e un dibattito che ha riguardato tutte le forze politiche, abbiamo messo ordine e dato una prospettiva accettabile per portare avanti questo tipo di iniziative, che sicuramente hanno un effetto positivo sulle imprese sulle imprese che lavorano in un settore strategico come quello edilizio. Abbiamo ottenuto l'esenzione per altri tre mesi della TOSAP: si tratta di uno dei nostri obiettivi ed è stato raggiunto.

nel comparto delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco e per le tutele legali nei confronti di questi servitori dello Stato, che noi dobbiamo ringraziare e rispettare e che hanno organici assolutamente inadeguati.

però fare i conti con la realtà che ci dice che, proprio in questi giorni e in queste ore, c'è una recrudescenza della pandemia molto preoccupante, nonostante l'Italia sia stata protagonista di una campagna vaccinale che, con la nascita del Governo Draghi e il lavoro del generale Figliuolo, ha segnato un'evoluzione e un cambio di passo rispetto al passato. Siamo convinti che questa campagna sia stata fondamentale per far sì che quest'anno, a settembre, ottobre e novembre, non abbiamo dovuto assistere alla chiusura delle nostre attività. Come abbiamo visto, abbiamo garantito il lavoro per tutti gli operatori economici e la libertà di movimento per i nostri cittadini. Rispetto a un anno fa molto è cambiato. Il vaccino non è la panacea di tutti i mali nei confronti della pandemia, ma sicuramente è stato in grado di arginare, limitare i danni della pandemia e permettere al nostro sistema economico di operare e ai nostri cittadini di lavorare liberamente. La recrudescenza, però, ci preoccupa; non vorremmo assistere nuovamente alla stagione delle chiusure. Non bisogna quindi abbassare la guardia, anche perché i conti dello Stato non potrebbero sostenere una nuova stagione di ristori e di sostegni a causa delle chiusure delle attività. Si chiude un anno in cui abbiamo fatto passi in avanti. Noi siamo convinti che la scelta della Lega di far parte di questo Governo sia stata una scommessa non facile. infatti all'interno di Governo in cui forze politiche molto diverse cercano di collaborare nell'interesse del Paese, ma, come ho detto, siamo convinti che sia stata una scelta giusta, perché molti dei risultati che abbiamo raggiunto anche in questa legge di bilancio rispecchiano la nostra impostazione. Senza la Lega al Governo probabilmente il taglio delle tasse avrebbe preso altre direzioni. del nostro movimento di far parte di un Governo così eterogeneo è ampiamente ripagato, perché siamo convinti che abbiamo fatto l'interesse dei cittadini. un'ultima preoccupazione, che è quella delle cartelle esattoriali. Su questo punto non siamo stati in grado, purtroppo, di dare risposte ai cittadini che sono ancora in grave difficoltà; non a cittadini che non vogliono pagare le tasse, ma a cittadini che non sono in grado di pagarle. Non c'è stata una risposta adeguata su questo tema, nonostante i nostri sforzi, i nostri tentativi. Il rinvio non è la risposta. Servono operazioni operazioni più coraggiose di rottamazione delle cartelle, altrimenti si rischia di gettare nella disperazione troppe famiglie, di mettere fuori gioco troppe attività. Questo, credo, sarà l'impegno che dovremo affrontare il prossimo anno e la Lega sicuramente sarà protagonista in questa battaglia. *(Applausi)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori, di legge di bilancio 2022 è un intervento espansivo, nel solco di tutti i provvedimenti adottati durante il Governo Conte II, per far fronte alla crisi pandemica. una manovra che punta a soddisfare la forte domanda di beni pubblici, resa ancor più forte in questo drammatico tornante della nostra storia, di beni come lavoro, sanità, istruzione, ambiente, protezione sociale, attenzione per la casa. È un intervento espansivo, voglio sottolinearlo con forza, fortemente caratterizzato dalla misura che più di ogni altra sta generando un impatto positivo sul rilancio del Paese, sulla crescita del PIL, sulla generazione di posti di lavoro, sul conseguimento di obiettivi ambientali in termini di risparmio energetico. Mi riferisco al superbonus al 110 per cento, ideato dal MoVimento 5 Stelle e approvato dal Governo Conte II nel maggio del 2020. Non starò qui a fare l'elenco di tutti i centri di ricerca, le istituzioni pubbliche, gli osservatori che hanno certificato, numeri alla mano, il successo del superbonus. Mi permetto, semmai, di rilevare che non è vero che è solo a causa del superbonus che stanno crescendo i prezzi di alcuni materiali. Non è vero che solo il superbonus ha generato frodi per 4 miliardi Quanto al primo punto, contiamo che il Governo sappia che l'aumento dei prezzi di alcuni materiali sta contraddistinguendo molti altri Paesi europei, che certo non hanno il superbonus, ma che forse vorrebbero averlo, considerate le parole di elogio dei commissari Timmermans e Simson. Quanto al secondo punto, è doveroso spiegare bene che la stessa Agenzia delle entrate ha dovuto correggere il dato, spiegando che i 4 miliardi riguardano frodi rilevate a proposito di tutti i bonus edilizi ed energetici. Di più, quei 4 quei 4 miliardi fanno riferimento a crediti fiscali oggetto di attività di verifica, cosa ben diversa dal dire che sono tutti frutto di frode conclamata. Fatta questa necessaria precisazione, è un dato che anche con questa legge di bilancio il MoVimento 5 Stelle si conferma la forza politica più orientata alla tutela di quel bene così prezioso per gli italiani che è la casa. Con il superbonus, ma anche grazie alla conferma degli altri bonus edilizi, a proposito dei quali il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto il recupero del meccanismo della cedibilità dei crediti di imposta, stiamo proteggendo le case degli italiani, le stiamo migliorando, le stiamo rendendo più efficienti dal punto di vista energetico, ne stiamo aumentando il valore; all'interno di tale filosofia si inseriscono tutti i miglioramenti che, grazie a noi, sono stati apportati al superbonus e sono stati ampiamente discussi dai colleghi. anche altre novità introdotte dal Movimento 5 stelle, come il fondo per sostenere il *cohousing* per gli anziani soli. Certo, non è stato facile fare tutto questo, non è stato facile analizzare il disegno di legge di bilancio, che è arrivato solo a metà novembre qui al Senato. *(Applausi)*. Non è stato facile lavorare Non è stato facile lavorare sapendo che il MEF è stato impegnato fino a circa due settimane fa sul PNRR e non poteva analizzare i nostri emendamenti. Non è stato facile avere a disposizione un perimetro economico ristretto per dare finalizzazione a sacrosante proposte parlamentari. In sintesi, non è stato facile lavorare su questo disegno di legge in una condizione che definire di forte compressione dei tempi e delle prerogative parlamentari sarebbe un eufemismo. Ed è solo per il senso di responsabilità di tutti noi, di tutte le forze politiche, che oggi riusciamo a condurre in porto il disegno di legge di bilancio. Comunque, è corretto rilevare il meccanismo di lavoro che ha visto la creazione di tavoli condivisi tra Gruppi politici e Governo è stato in grado di farci arrivare a una sintesi condivisa su molti temi e i Gruppi politici qui presenti, tutti, hanno cooperato per arrivare al risultato. Ma nella manovra c'è tanto altro: c'è un intervento di abbassamento delle aliquote Irpef con contestuale riduzione del loro numero, come non se ne vedevano da tempo. Il risultato è un taglio consistente delle tasse che guarda al ceto medio, messo a dura prova dalla totale assenza di segnali negli anni, ma allo stesso tempo anche alle fasce reddituali più basse, peraltro già beneficiate l'anno scorso dalla riduzione del cuneo fiscale operata dal Governo Conte II. Sempre in tema fiscale, c'è lo storico azzeramento dell'IRAP su oltre 800.000 piccoli contribuenti, che dall'anno prossimo potranno finalmente fare a meno di un'imposta che ha sempre creato duplicazioni e difficoltà amministrative. Siamo riusciti a confermare altri importanti misure del Governo Conte II, prorogando per altri tre mesi l'esonero dal pagamento della TOSAP per esercizi pubblici come bar e ristoranti, tra i più penalizzati dalla crisi pandemica, abbiamo dato un ulteriore boccata d'ossigeno ai contribuenti, portando da due a sei mesi il tempo per pagare le cartelle esattoriali che saranno notificate nei primi tre mesi dell'anno prossimo. di legge abbiamo difeso e potenziato, con un altro miliardo di euro, il reddito di cittadinanza, che tanta importanza ha rivestito nello stendere una rete di protezione intorno a categorie fragili, come bambini, disabili e anziani, che senza questo strumento avrebbero pagato un prezzo altissimo di fronte al Covid. Il reddito di cittadinanza è stato elogiato, anche negli ultimi mesi, da tutti i principali organismi che si occupano di povertà, dalla Caritas a Save the Children, alla Comunità di Sant'Egidio. La Caritas, per esempio, ha definito la misura uno «strumento Con la manovra approntiamo una risposta anche a beneficio di famiglie e imprese messe alle strette dal rincaro delle bollette, innescato dall'aumento del costo dell'energia. I fondi nel testo finale sono quasi raddoppiati, fino a 4 miliardi, il tutto in attesa di una riforma complessiva del sistema delle bollette, che nella nostra proposta deve portare ad abbattere strutturalmente i costi. Su questo, come su altri temi, considerando che non siamo ancora fuori dalla pandemia, dobbiamo essere pronti a stanziare più risorse il prossimo anno. Dobbiamo essere pronti a un ulteriore scostamento di bilancio, perché per noi aiutare una famiglia di anziani, aiutare una mamma o un papà con un figlio disabile, aiutare chi è rimasto senza lavoro, era, è e sarà sempre debito buono. Per la sanità ci sono 4 miliardi in più per potenziare il Fondo sanitario nazionale e sostenere la fase di contrasto alla pandemia con un intervento che, nella scia di quanto fatto dai Governi Conte, finalmente inverte quell'odioso *trend* di definanziamento della sanità che ha prodotto effetti tanto negativi, resi drammaticamente chiari dall'esplosione della pandemia. Siamo riusciti a rendere triennale il nostro piano Transizione 4.0 per incentivare le imprese nella transizione verde e digitale, abbiamo aumentato i fondi per il nostro *export*, che grazie alle nostre misure sta mettendo a segno un anno da *record*. L'Italia sta imboccando una strada di rilancio testimoniata dalla forte crescita che l'economia registrerà quest'anno, con un PIL ormai dato da tutti gli osservatori a oltre +6 per Il merito è tutto delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, delle nostre famiglie, della resilienza di un Paese che ha saputo resistere e rialzarsi. La manovra 2022 intende premiare questo sforzo cercando di fornire tutti gli strumenti per consolidare gli effetti positivi che stiamo vedendo.

Io sospenderei non per mezz'ora, come ha chiesto il presidente Pesco, ma per cinque minuti, invitando il Presidente a venire in Aula a riferire. La seduta è sospesa.

ritardo "a spizzichi e bocconi". l'abbiamo studiata in Commissione, su questa sono state fatte delle scelte e queste scelte, per essere tradotte in un parere, hanno bisogno di tempo. Quindi, serve ancora mezz'ora. siamo in grado di non far stare qui tutti in attesa e di prevedere un tempo ragionevolmente vicino al giusto, o se ogni mezz'ora avete bisogno di più tempo.

oggi pomeriggio. Tutte le previsioni fatte oggi sono state disattese, andiamo avanti con rinvii di mezz'ora, un'ora, venti minuti, mezz'ora.

perché praticamente non ci ha detto niente. Non credo che, per la dignità di ogni componente di questa Assemblea, si possa essere ostaggio; per cui va bene tutto, ma la pazienza ha dei limiti. Vogliamo sapere, Presidente, qual è il prosieguo della nottata. Ci è consentito o non è democratico fare questa domanda alla Presidenza? Vogliamo sapere fin quando ritenete di tenerci in ostaggio qua dentro senza dirci niente, Grazie

Avviserò la Presidente della richiesta di Fratelli d'Italia, perché comporterebbe la necessità di una Capigruppo. Facciamo nel

Il Natale lo si può fare dovunque. Ci sono altri interventi oltre a questo brillante?

e anche le condizioni sulle osservazioni: sia le osservazioni sulle osservazioni, che le condizioni. Per il Governo il parere va bene e, quindi, anche le osservazioni saranno inserite nel testo del maxiemendamento.

se la forma e sostanza e la forma è l'umiliazione del Parlamento, allora la sostanza è l'umiliazione delle categorie produttive. Oggi con il PNRR avete intrappolato l'Italia, consegnandola alla globalizzazione finanziaria. Oggi avete cominciato anche a distruggere il comparto della balneazione, montando ad arte la commedia delle gare e delle aste, facendo leva sui canoni di concessione troppo bassi. Bastava adeguarli, ma voi volete regalare le nostre spiagge ai grandi gruppi. Le concessioni non le toccate quando - per esempio -c'è il *business* delle acque minerali, con altissimi profitti e bassissimi canoni. Che dire dei soldi che avete regalato di fatto ai Benetton, ad Atlantia? Vergognatevi! Parlate del caro bollette luce e gas, ma non fate nulla, perché le micro-imprese e le PMI pagheranno, al netto del "bla bla bla", bollette carissime e voi non inciderete per niente. Puntate sul superbonus dell'edilizia, ma non vi accorgete che nella filiera stanno saltando piccole e medie imprese, per le cartelle esattoriali, per il DURC, per le banche. Il superbonus batterà in testa, perché le materie prime costano sempre di più e c'è anche scarsità delle stesse e questo metterà in difficoltà una buona idea. Questa manovra è caotica, come il metodo che l'ha portata qui. Voi siete, del resto, maestri della confusione. Volevate salvare il Natale: state mettendo in *lockdown* leggero. Le farmacie sono prese d'assalto. Sui *green pass* c'è grande confusione, regna il *caos* sulla durata dei sieri. Insomma, più che una manovra, mi sembra un altro inganno ai danni degli italiani.

Mantero).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mantero.

La 5a Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi

una nuova finestra") Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della prima sezione. Tale Nota è stata deferita alla 5a Commissione permanente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5a Commissione permanente in ordine alla Nota di variazioni. *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 è stata predisposta al fine di recepire nel disegno di legge di bilancio, da un lato, gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica e, dall'altro, gli effetti che si sono prodotti a seguito della conversione nella legge n. 215 del decreto-legge n.146 del 2021. In relazione a quanto precede, la presente Nota aggiorna i valori contabili dell'*ex* articolo 216, «Totale generale della spesa», del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2022-2024 in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione dell'entrata, tabella n.1, e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri, tabelle da 2 a 16. Si producono in conseguenza anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli. I prospetti sono organizzati per unità di voto e gli allegati tecnici per capitoli presentano l'intero bilancio dello Stato, con evidenza delle unità e dei capitoli che hanno subito variazioni, per effetto degli emendamenti al disegno di legge. Le variazioni connesse agli emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne, distintamente per la sezione 1 e la sezione 2. *(Applausi)*. Mai una Nota di variazioni fu così applaudita. Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni. Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura,